grazie a tutto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

Il relatore, senatore Dell'Olio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) è uno degli strumenti fondamentali del ciclo della programmazione economica e finanziaria del Paese. Fra i contenuti principali della NADEF ci sono, in particolare, l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche di finanza pubbliche, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal Documento di economia e finanza, le eventuali modifiche ed integrazioni al DEF, conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al programma di stabilità e al programma nazionale di riforma, l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale, l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo e l'indicazione di disegni di legge collegati. Alla NADEF, inoltre, è annessa la relazione al Parlamento di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, sull'aggiornamento del piano di rientro. Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, la NADEF 2020 riporta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso, figlia della nota contrazione del sistema economico a causa della pandemia. Cercherò di limitare, per quanto possibile, l'utilizzo di numeri e percentuali in questo discorso, rimanendo sul lato fattuale del quadro storico che attesta tale situazione. Nonostante gli interventi messi in atto dai vari Governi e le misure di politica monetaria introdotte dalle banche centrali, c'è stato un blocco generale del commercio mondiale, che si è accentuato nel secondo trimestre 2020 e ha interessato tutte le principali economie avanzate, incluse quelle di Stati Uniti e Cina. Se, oltretutto, consideriamo che l'Italia aveva da tempo delegata la capacità produttiva a tali Stati esteri per l'approvvigionamento, non solo di materie prime, ma anche di prodotti finiti (mi riferisco, ad esempio, a tutti i presidi sanitari per i quali abbiamo avuto scarsità di approvvigionamento durante la prima fase del *lockdown*) e la conseguente riduzione di fornitura dovuta a un maggiore consumo interno di tali Paesi, ci si può facilmente rendere conto dell'impatto negativo che si è avuto nel nostro Paese. Il profilo macroeconomico si complica se si considera il potenziale aumento del prezzo del petrolio. Da un minimo storico di 20 dollari al barile nella prima fase della pandemia, rispetto ai 60 di fine febbraio, si manifestano segnali di ripresa che hanno portato il prezzo già a 40 dollari al barile. Il profilo di rischio sottolineato dalla NADEF è coerente con le valutazioni espresse dai principali istituti previsori, fra cui OCSE, FMI, Eurostat e BCE, segno che la stessa è stata redatta in maniera prudente e coerente con la fase storica che stiamo vivendo, senza prevedere possibilità di riprese che siano estremamente ottimistiche e non realistiche, distanti dalla realtà. In tutto questo, comunque, è corretto riportare che si è registrata una generale e graduale ripresa, a partire dai mesi di maggio e giugno, con il riavvio delle attività produttive, ma con un andamento disomogeneo fra i vari Paesi. Una nota particolare in merito al commercio con l'estero. Sebbene nei primi due mesi dell'anno il livello delle esportazioni si fosse mantenuto con tassi di crescita positiva, gli effetti della pandemia si sono riversati anche sulle esportazioni, specie nei confronti dei mercati extra UE, penalizzando di più la Cina rispetto agli Stati Uniti. Adesso i flussi commerciali sono in ripresa, a partire da luglio, andando a colmare il *gap* che si era creato in particolare verso i mercati extra Unione europea. Siamo però realisti: nonostante questi miglioramenti, l'attività economica del 2020 resterà significativamente al di sotto dei livelli del 2019. Ciononostante, il livello degli indici di fiducia valutati dall'Istat il Paese sta apprezzando quanto è stato fatto dal Governo in questa delicata e soprattutto assolutamente inaspettata situazione. La NADEF presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico. Per quanto riguarda il profilo tendenziale, la ripresa dell'economia è fortemente influenzata dall'andamento della domanda, che risente ancora dell'impatto della crisi. È per questo che la NADEF

del DEF), a causa della previsione dell'impatto espansivo sulla crescita che verrà generato dalle misure di politica fiscale introdotte a maggio e ad agosto. La nuova previsione, inoltre, considera anche l'ipotesi di una gestione controllata dei focolai, che consentirà di non arrivare a un *lockdown* a livello nazionale, l'arrivo dei vaccini anti Covid-19 entro il primo trimestre del 2021 e una loro distribuzione su larga scala. Con questa ipotesi di base si prevede che si possa ritornare a un PIL pre-crisi nel 2023. Come è noto, l'Ufficio parlamentare di bilancio si deve esprimere sulla NADEF e in questo caso l'ha fatto con una lettera del 21 settembre, in cui ha validato queste previsioni, pur sottolineando la presenza di significativi rischi al ribasso sulla crescita reale del PIL. Il mercato del lavoro ha subìto una contrazione significativa nel 2020. L'intervento del Governo però, con le misure di estensione della possibilità di ricorso alla cassa integrazione e il divieto di licenziamento, hanno determinato una tenuta dei livelli occupazionali, portando la stima di riduzione dell'occupazione complessiva all'1,9 per cento su base annua. Si tenga presente che tale valore, riferito al secondo trimestre 2020 (sempre su base annua), era pari al 3,6 per cento; quindi l'impatto delle misure messe in atto è stato efficace. Secondo gli ultimi dati Istat (ottobre 2020) ad agosto continua però la crescita dell'occupazione, con una percentuale molto più forte fra i minori di trentacinque anni. Dal punto di vista del quadro macroeconomico programmatico, la NADEF tiene conto degli interventi straordinari per il sostegno e il rilancio dell'economia che il Governo intende portare avanti col PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), nell'ambito della procedura per l'accesso ai fondi stanziati con il programma Next generation EU, dotato di 750 miliardi di euro nel periodo 2021-2027. La manovra di finanza pubblica per il 2021-2023 punterà a sostenere la ripresa dell'economia, con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021, che si andrà riducendo nel 2022, per poi puntare a un significativo miglioramento del saldo di bilancio nel 2023. I principali obiettivi della politica di bilancio possono essere così riassunti. A breve, sostenere i lavoratori e i settori produttivi più colpiti dalla pandemia, fintanto che perdurerà la crisi da Covid-19. Poi, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, valorizzare appieno le risorse messe a disposizione dal Next generation EU per realizzare un ampio programma di investimenti e riforme, di portata e profondità tali da portare l'economia su un sentiero di crescita sostenuta ed equilibrata. Rafforzare gli interventi a sostegno della ripresa nel Mezzogiorno e nelle aree interne, per migliorare la coesione territoriale ed evitare che la crisi da Covid-19 accentui le disparità fra le diverse aree del Paese. Attuare un'ampia riforma fiscale che migliori l'equità, l'efficienza e la trasparenza del sistema tributario, riducendo anche il carico fiscale sui redditi medio-bassi, coordinandola con l'introduzione di un assegno unico universale per i figli. Assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse verso gli utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini e dell'equità e della produttività dell'economia, ipotizzando che la crisi sia gradualmente superata nei prossimi due anni. Ricondurre l'indebitamento netto della pubblica amministrazione verso livelli compatibili con una continua e significativa riduzione del rapporto debito-PIL. In termini di ambiti principali, nella Nota si prevedono il rifinanziamento delle cosiddette politiche invariate non coperte dalla legislazione vigente (per esempio missioni di pace, rifinanziamenti di alcuni fondi d'investimento, fondo crisi d'impresa); il completamento del finanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente (i cosiddetti 100 euro); il finanziamento del taglio contributivo al Sud, già introdotto dal decreto-legge agosto, limitatamente alla seconda metà del 2020;

per incrementare gli investimenti pubblici e aumentare le risorse per la ricerca, formazione, digitalizzazione e riconversione dell'economia in chiave di sostenibilità ambientale. Il nuovo obiettivo programmatico del 2021 risulta pertanto superiore rispetto al livello di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento con approvazione dell'ultima relazione del 22 luglio.

2020 reca altresì l'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023, in particolare per il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio periodo. Infatti, l'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che eventuali scostamenti temporali dal saldo strutturale e dall'obiettivo programmatico siano consentiti in caso di eventi eccezionali e previa autorizzazione approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti, indicando nel contempo il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine. Il comma 5 stabilisce anche che il piano di rientro possa essere aggiornato al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali, ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Si ricorda che la Commissione europea ha deciso l'applicazione della cosiddetta *general escape clause* per l'anno in corso per assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra nell'ambito del proprio bilancio per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l'emergenza epidemica e delle misure per contrastare gli effetti recessivi sull'economia europea della diffusione del Covid-19. Questo permette agli Stati di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento, ma non sospende l'applicazione del patto di stabilità e crescita né le procedure del semestre europeo in materia di sorveglianza fiscale. Gli obiettivi dell'indebitamento netto sono fissati pertanto a -7 per cento nel 2021, -4,7 per cento del 2022 e -3 per cento nel 2023. Per gli anni seguenti si prefigura un ulteriore significativo miglioramento del saldo di bilancio, tale da assicurare una riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL in tutti gli anni della previsione.

per l'anno 2019 la regola del debito non viene rispettata in nessuna delle tre configurazioni definite dal patto di stabilità e crescita; sulla scorta delle previsioni, il Governo sostiene che la regola non la rispetterà neanche per 2020 a causa della crisi economica conseguente alla pandemia. Il rapporto debito-PIL programmatico del 2020 sarà superiore di circa 30 punti percentuali rispetto alla soglia del criterio retrospettivo, di 12,3 punti rispetto alla soglia di quello prospettico e di 15 punti rispetto alla soglia determinata dal criterio del debito corretto per il ciclo. La NADEF pertanto conferma l'approccio già avanzato nel DEF, volto a ridurre il rapporto debito-PIL verso la media dei Paesi dell'area euro nel prossimo decennio, attraverso una strategia basata sul conseguimento di avanzi primari di bilancio in un contesto di rilancio degli investimenti pubblici e privati, ottenuto anche con le risorse dello strumento europeo Next generation EU, i cui effetti non sono tuttavia, per motivi prudenziali, incorporati nelle stime della finanza pubblica. ad intervenire. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 5, della legge n. 243 del 2012, la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo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

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, membri del Governo, per valutare in maniera adeguata la Nota di aggiornamento al DEF ora più che mai non si può prescindere dal contesto, sia generale sia politico, in cui stiamo vivendo. A livello generale, è di tutta evidenza che il prossimo anno - e forse anche i successivi - sarà caratterizzato dall'andamento della pandemia da coronavirus sia a livello mondiale che a livello nazionale, con tutte le conseguenze sanitarie, sociali ed economiche che questo implica. Dal punto di vista politico, in Italia risulta chiaro come la pandemia sia diventata anche un alibi con cui l'Esecutivo, per far fronte alla propria debolezza politica,

ottimismo che il ministro Gualtieri ha manifestato pubblicamente in più occasioni. L'Ufficio parlamentare di bilancio, se avalla seppure con criticità il rimbalzo del 2021, non approva però le previsioni per il biennio successivo. D'altronde, secondo l'OCSE, sulle prospettive di ripresa globali persiste ancora una considerevole incertezza legata all'evolversi della pandemia, per cui una recrudescenza del virus o misure di contenimento più rigorose potrebbero portare ad una riduzione della crescita del PIL globale, con una disoccupazione più elevata e un periodo più prolungato di investimenti deboli. Nella NADEF si tiene conto dello sviluppo della pandemia, ma si tiene anche conto della possibilità di avere un vaccino a disposizione già in primavera, cosa che tutti ci auguriamo ma che non è per nulla scontata. Su questo quadro si innestano le politiche e le riforme che il Governo va ad attuare. La proroga dello stato di emergenza, le misure di restrizione adottate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche tutti gli innumerevoli annunci che infieriscono psicologicamente sugli imprenditori e sui consumatori influiscono negativamente sugli andamenti dell'economia e mettono in discussione le previsioni del Governo. Quello che emerge dalla NADEF è che l'Esecutivo, in attesa dei fondi europei che non si sa quando verranno e a fronte della scelta di non accedere al MES, ha bisogno impellente di reperire risorse per poter proseguire le proprie politiche sostanzialmente assistenzialiste. Su che cosa ci si basa? Solo ed esclusivamente sul recupero dell'evasione fiscale. Già partite ben 9 milioni di cartelle esattoriali, il 90 per cento delle quali - è già stato ricordato - sotto i 5.000 euro. Ma vi sembra tutto sommerso? Possibile che si senta solo parlare di recupero dell'evasione, identificandolo esclusivamente con il sommerso, e che non si senta mai - ripeto, mai - che il Governo imponga alla pubblica amministrazione di saldare i propri debiti commerciali nei confronti delle imprese stimati attualmente in circa 53 miliardi di euro? Il paradosso arriva al culmine quando si legge nella NADEF che verrà istituito un fondo dove confluiranno i proventi recuperati dall'evasione, le maggiori entrate per la minore decontribuzione, le tasse dell'industria della plastica e gli effetti della *compliance* del contribuente. Con questo fondo sarà finanziata la riforma fiscale. Della serie: pagare sicuramente di più adesso per forse pagare meno poi. Un'assurdità. Consideriamo poi che l'ammontare dell'evasione, stimata in più di 110 miliardi, è almeno pari - e da alcuni valutata ben inferiore - al costo della burocrazia. Ma il Governo anche nel provvedimento in discussione non fa nessun accenno ad alcun intervento veramente significativo di sburocratizzazione. I costi della cattiva burocrazia e i mancati pagamenti della pubblica amministrazione costano alle imprese - questo dobbiamo ricordarlo -, secondo una stima della CGIA di Mestre, circa 100 miliardi all'anno. *(Applausi)*. A conferma di quanto detto, una delle tante riforme attese ed annunciata sia dal presidente Conte che dal ministro Gualtieri, la riforma fiscale, è proposta come legge delega, ma tutti conosciamo i tempi biblici di tale provvedimento e i decreti legislativi che implica; altro che pronta a breve: ci vorranno anni. È evidente che intervenire sulla revisione del sistema fiscale, sullo snellimento e sulla riduzione delle tasse che incidono per il 48,2 per cento non è proprio nelle priorità di questo Governo. Per le imprese non si fa proprio nulla, e ricordiamo che la diminuzione del cuneo fiscale è solo per per i lavoratori dipendenti. I commercialisti hanno lamentato - proprio in questi giorni - che, esattamente un anno fa, insieme a Confindustria, avevano presentato al legislatore e all'amministrazione finanziaria un corposo documento con le proposte di semplificazione fiscale e di riforma del sistema tributario del Paese. E poi? Nessun cenno di riscontro in merito. Quindi, il Governo non solo non ascolta l'opposizione, ma neppure chi, in questo Paese, in forza della propria attività, diventa portatore di interessi diffusi. hanno dovuto minacciare uno sciopero per riuscire a far spostare la scadenza del pagamento delle imposte ai fini IRPEF e IRES, e si sono dovuti accontentare della proroga solo per i soggetti ISA e i forfettari, in un momento di crisi pazzesca in cui il Governo ha obbligato le imprese a chiudere, perché il *lockdown* - lo dobbiamo ricordare - è stata un'imposizione del Governo. Lo stesso Governo non solo non ha bloccato il pagamento delle imposte, ma addirittura non ne ha spostato la scadenza. Ebbene, gli italiani non hanno bisogno di tutto ciò; hanno necessità

e a generare posti di lavoro. Ora la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti hanno dato sollievo a milioni di lavoratori, ma non hanno risolto problema; l'hanno solo spostato. I fondi del SURE sapranno dare ancora un po' più di ossigeno, ma, ripeto, ma, ripeto, il problema bisogna risolverlo alla radice. E non pensiate sia sufficiente realizzare solo qualche infrastruttura per far ripartire un Paese. L'ha ben detto il presidente di Société générale, Lorenzo Bini Smaghi, quando avverte che gli investimenti, se non sono supportati da vere riforme, resteranno opere sterili. Non vorremmo che anche in questo caso i provvedimenti collegati al bilancio previsti nel documento restino lettera morta, con centinaia e centinaia di decreti attuativi che latitano nei Ministeri; che a forza di libri dei sogni questi non si trasformino in incubi per il Paese, perché, prima o poi, gli italiani si sveglieranno.

Presidente, vice ministro Misiani, colleghi, la NADEF, con lo scostamento che ci apprestiamo a votare, rappresenta una strategia abbastanza organica. Qualche economista la definisce plausibile; a me piace di più definirla coerente, perché dà una buona visione di un mix di prospettiva (anche molto equilibrato) e prudenza, perché le stime fatte in più punti sottovalutano gli effetti positivi sia delle entrate sia delle ricadute in termini positivi sulle basi imponibili, quindi in termini di PIL, di tutte le manovre espansive che, anche grazie al Next generation EU, ci apprestiamo a inserire nel nostro contesto di bilancio nazionale. È evidente che la NADEF cerca di puntare l'accento sulla fase positiva, espansiva delle politiche in prospettiva; parla moltissimo delle politiche che ci apprestiamo a introdurre grazie allo stimolo europeo, quindi alle grandi transizioni europee e nazionali che ci aspettiamo, e anche al grande piano di coesione nazionale e territoriale

Tutto questo viene fatto in un quadro economico coerente e credibile. Quanto al quadro macroeconomico, è evidente che il PIL presenta una flessione molto forte, perché - 9 per cento è un valore che può anche spaventare. È un PIL tuttavia meno negativo rispetto alle previsioni di qualche mese fa, continua a essere leggermente positivo rispetto alle previsioni internazionali. Ieri abbiamo infatti visto il Fondo monetario internazionale prevedere per l'Italia un calo

È evidente che moltissima parte dei dati macroeconomici dipende dalla pandemia: la stiamo gestendo meglio di altri, ma

avremo ovviamente ulteriori aggiustamenti e ulteriori valutazioni da fare. Per quanto riguarda invece il percorso di finanza pubblica e quindi la nostra politica

che appoggiano la presidenza von der Leyen e appartengono al Partito popolare europeo. Il Partito popolare a livello europeo ha infatti condiviso queste strategie, che appartengono allo scostamento, che oggi ci apprestiamo a votare. Per quanto riguarda la spesa per interessi, continuando a parlare del percorso di finanza pubblica, beneficia di tutte le politiche monetarie espansive.

l'andamento del *deficit*. Abbiamo visto disavanzi primari negativi in tutte le grandi crisi dal 1975, al 1991, fino al 2009, questo non può non impegnarci per il ritorno ad un equilibrio, che ci aspettiamo però solo verso il 2023. Il rapporto tra debito e PIL aumenta di 23 punti nel 2020, nel 2020, per supportare le politiche espansive. Il debito pubblico resta sostenibile: tutti i previsori e tutti i valutatori l'hanno confermato.

è la prospettiva, che leggiamo nello scostamento e in quello che vorremo fare poi, nella prossima legge di bilancio, con questo ulteriore scostamento. Rispetto all'obiettivo di medio termine, il *deficit* si è spostato dal suo sentiero di 8,6 punti percentuali. Per ogni punto percentuale di PIL, il *deficit* è aumentato di 0,9 punti. Quindi stiamo parlando di una situazione grazie a tutto *general escape clause* e con la disapplicazione parziale del Patto di stabilità e crescita. Ancora una volta, quindi, invito i colleghi che fanno parte di questa cultura politica a fare una valutazione sul prossimo voto sullo scostamento.

a quanto leggiamo nella NADEF, il recepimento delle politiche europee del Next generation EU è molto prudente: nella prima fase vi sarà un assorbimento molto forte delle sovvenzioni, e cioè dei contributi a fondo perduto che non dovremo restituire, mentre dal 2024 in poi - quindi nel 2024, nel 2025 e nel 2026 - si riequilibrerà con una maggiore presenza dell'indebitamento e, quindi, del ricorso ai prestiti europei che sono ovviamente da rimborsare, come tutti i prestiti del resto, ma a tassi particolarmente agevolati.

quasi 38 miliardi, di cui 24 di indebitamento (13 di indebitamento nazionale e 11 di indebitamento europeo) e 14 di sovvenzioni

È molto importante e secondo me la legge di bilancio dovrà portare molto con sé del *new normal*. Mi riferisco - ad esempio - ad alcuni temi specifici: lo *smart working*, così com'è, è un *home working* e non porterà allo stimolo che ci aspettiamo.

e anche nei rapporti interpersonali - lo abbiamo sentito pure ieri in quest'Aula nelle parole degli esponenti della maggioranza e dal presidente Conte - ci sono stati rivolti reiterati appelli alla collaborazione e al senso di responsabilità. Ebbene, siccome non siamo abituati a farci accusare ingiustamente, ci tengo a chiarire che fare appelli alla responsabilità in questo contesto, nel modo in cui avete operato, è un po' come, signor Presidente e caro viceministro Misiani, invitare a costruire assieme una casa il giorno prima dell'inaugurazione. Voi, a pochi minuti dall'approvazione in Aula della Nota di aggiornamento al DEF, pretendereste senso di responsabilità dall'opposizione. ritengo che siamo davvero vicino al ridicolo o alla presa in giro. Se davvero la maggioranza intenderà collaborare con l'opposizione, non ce lo dica più di un provvedimento, ma ce lo venga a dire con i tempi dovuti, in modo tale che davvero si possa costruire assieme un percorso nell'interesse del Paese. Ciò detto e chiarito - spero mi sento in dovere di ringraziare i tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze per l'opera di assemblaggio che, come sempre, hanno fatto in modo magistrale; modo magistrale; meno mi sento di ringraziare, invece, la maggioranza e il Governo per i contenuti che improntano la Nota di aggiornamento al

schiettamente pre-elettorale». In sostanza, dice quello che noi affermiamo da mesi: tutti i provvedimenti che state prendendo sono, nella migliore delle ipotesi, degli analgesici, che non hanno davvero a cuore le sorti del Paese. Sto citando, peraltro, non esponenti della mia cultura politica, ma esponenti sinceri intellettualmente corretti della vostra parte politica.

dopo di voi. Vi state semplicemente adoperando per creare misure di consenso e ho ragione, quindi, di temere che anche l'utilizzo dei fondi europei - e poi mi soffermerò su questo - seguirà la stessa logica elettoralistica e a breve termine, con la differenza che, se la politica a breve termine nel passato ha portato il Paese alle attuali condizioni, l'utilizzo di una logica a breve termine con risorse straordinarie - come saranno i 200 miliardi di

Non c'è un'assoluta discontinuità nella lettura della NADEF tra il presente e il futuro. In un momento eccezionale quale quello era necessaria una netta discontinuità; una discontinuità nei numeri e una discontinuità dei progetti. Se non si trasforma il Paese in un momento eccezionale come questo, quando lo vogliamo fare? fare? Accanto al tema del risanamento dei conti pubblici che caratterizzano questa manovra in senso elettorale, anche le fonti destano preoccupazione. Le fonti su cui si fonda una buona parte dell'impostazione contabile della NADEF derivano dal *recovery fund*.

Ecco un altro aspetto che rende - come ha detto una collega di Forza Italia - le fonti ballerine all'interno della Nota dovuto invece prevedere, a livello di contenuti e di strategia, il Documento di programmazione economica? Come peraltro la stessa maggioranza aveva fatto trapelare nei momenti antecedenti

Possiamo vedere che tutta la stampa specializzata - e non certo i giornali di propaganda di una parte o dell'altra, - ma, ad esempio, lo stesso «Il Sole 24 Ore» caratterizza in modo chiaro che nella NADEF, al di là di vuote parole, non c'è nulla che rispecchia la riforma fiscale, come non c'è nulla - e lo abbiamo visto ieri - nel Piano di ripresa e di resilienza

si parla unicamente di cuneo fiscale sul lavoro dipendente. Per questa maggioranza la ripresa del Paese, la ripresa degli investimenti e la crescita del PIL si attueranno solamente con la riduzione del cuneo fiscale, che peraltro è coerente

che la prospettiva fondamentale è ridurre il carico fiscale sui redditi bassi, vorrei ricordare al ministro Gualtieri che un italiano su quattro non paga imposte e che il 41 per cento dei dichiaranti pagano oltre il 90 per cento dell'IRPEF. In sostanza, vorrei dire che, dal combinato disposto degli 80 euro e poi dei 100 euro, oggi di fatto le imposte pagate da coloro che arrivano alla soglia dei 40.000 euro sono pressoché zero. Quindi, al di là del populismo e della demagogia, dobbiamo invece dire un'altra cosa e, cioè, che la ripresa del Paese e l'utilizzo della leva fiscale andranno fatti in una direzione completamente diversa, ovvero nella direzione dell'impresa e delle aziende. Noi dobbiamo riportare capitali nelle imprese; dobbiamo rendere conveniente agli stranieri investire nel nostro Paese, ma anche agli italiani stessi e, quindi, dobbiamo incentivare l'impresa con la leva fiscale. Dobbiamo riportare ricchezza. Altro che misure populiste! Mi dispiace dovermi riferire al collega Monti

facendo riferimento alla revisione della spesa pubblica e alla ristrutturazione della pubblica amministrazione, che tutti a parole indichiamo come uno dei capisaldi capisaldi che servirebbe alla ripresa del Paese. Allora perché nella NADEF non è riportato alcunché e non sono riportati i costi sociali di una ristrutturazione della pubblica amministrazione? Non ve lo potete permettere e perché guardate solamente alle prossime elezioni politiche, con le quali già saprete che gli italiani

Concludo con il tema del credito. Nella scorsa legislatura per salvare le banche avete distrutto il credito, il credito del territorio, le banche popolari, le casse rurali e oggi tutti, anche i presidenti di quella Cassa centrale banca che avete provveduto a costruire, dicono che non si può andare avanti così, che non sono più in grado di fare credito alle PMI. Nei territori gli sportelli stanno chiudendo e l'Unione dei Comuni montani lancia un grido di dolore in questa direzione. Voi cosa fate e cosa prevedete per la controriforma del credito e per ridare fiato al credito delle nostre banche? Non prevedete un bel niente e così oggi ci troviamo un sistema bancario la cui attività principale sono gli investimenti e le attività assicurative e non il credito all'impresa che deve fare ripartire il PIL.

Signor Presidente, signor Vice Ministro, desidero fare qualche considerazione sulla NADEF, che è oggetto del nostro dibattito, e vorrei esordire con un con un riferimento che non mi capita spesso di fare; un riferimento cioè di condivisione su quanto ha detto il senatore De Bertoldi. egli ha detto che ha l'impressione - chiedo scusa al collega se forse le parole non sono quelle letteralmente da lui usate che in questa fase della politica economica italiana e nell'opinione pubblica italiana ci sia un'eccessiva dipendenza da qualche cosa che si dà per scontato - il *recovery fund* e le sue immani benedizioni finanziarie - quando il percorso di quella costruzione politico economica europea è ancora abbastanza accidentato. Mi permetto invece di respingere con garbo al collega mittente quello che con superficialità rimarchevole ha detto in ordine alle manovre del 2011-2012, che possono essere condivise o no; ci possono essere state componenti anche rivolte a persuadere l'opinione pubblica che

e quella di Montecitorio hanno dato prova di grande responsabilità, accollandosi oneri di impopolarità politica che hanno contribuito per un intero anno a evitare che il Paese cadesse nel dissesto finanziario. italiani dicono che quell'austerità sia stata in fondo la vera causa della nascita del populismo.

qualche provvedimento di forte restrizione. No, è venuto dal fatto che i partiti tradizionali, quelli ai quali sono ancora grato perché hanno sostenuto per un anno l'onere di risanamento del Paese - e vanno dal a Forza Italia, a Fratelli d'Italia (perché, senatore De Bertoldi, non eravate ancora nati, ma facevate parte delle forze che hanno sostenuto quelle operazioni che ora criticate aspramente), oltre, naturalmente, al centro - dopo un anno di responsabilità, semplicemente perché si avvicina... Sono sicuro che era un'osservazione interessante, ma purtroppo non l'ho sentita, ma ci sarà modo.

di una gigantesca propaganda ai populisti.

ma non dà veramente l'impressione che bisognerebbe cercare di dare al Paese in questo momento, in cui siamo per un ripensamento dell'Europa per il disastro del Covid e per la buona gestione che il Governo ha fatto, per quanto ha potuto, sia del Covid,

costume politico, ma anche nell'opinione pubblica italiana l'idea che adesso i tempi sono veramente cambiati - e sono cambiati in peggio perché abbiamo dei problemi in più ma il fatto che il nostro Paese sia squilibrato tra la produzione delle risorse e l'uso delle risorse rimane. Il fatto che continuiamo, con maggiore o minore disinvoltura, a mettere enormi oneri a carico dei nostri figli e nipoti rimane. Ecco, quindi, che ci vorrebbe, anche nella gestione di breve periodo, un rigore particolare. In altri termini, se mi si dovesse chiedere qual è la mia più grande speranza per l'economia italiana nei prossimi tempi, io direi il *recovery fund*; e se mi si chiedesse qual è la mia principale preoccupazione, io direi il *recovery fund*, perché ha un effetto psicologico che viene prima e supera in velocità le resistenze polacche, ungheresi e dei Paesi frugali, eccetera. Già l'abbiamo incorporato trionfiamo per il fatto che noi siamo stati capaci di far cambiare una pagina storica all'Europa, mentre l'Europa, finalmente, dopo gli sforzi di tanti Governi - italiano, francese, spagnolo, eccetera - ha visto nella Germania un punto di cambiamento fondamentale grazie alla cancelliera Merkel. Ma l'Europa, che è basata su regole perché è una costruzione giuridica e non puramente della fantasia e del sogno (come qualche volta ci piacerebbe), dovrà reintrodurre regole sugli aiuti di Stato, anche perché - altrimenti - le imprese tedesche si mangerebbero tutte le altre, dato il volume di disponibilità finanziaria dello Stato tedesco. L'Europa dovrà reintrodurre - speriamo non in quella forma molto criticabile e criticata - un Patto di stabilità. La Banca centrale europea, come tutte le come tutte le banche centrali del mondo, passata questa fase, che speriamo passi, si appresta già a riconsiderare che il ruolo proprio e delle banche centrali in generale non è necessariamente - come si pensa in certi settori di questa finanziare con prodigi illimitati qualsiasi disavanzo dei Governi. Lo stesso ragionamento, quindi, varrà a proposito dello scostamento di bilancio, quella legge costituzionale che fu approvata nel 2012, con una tale maggioranza in Parlamento, superiore ai due terzi, da non dare luogo a *referendum* confermativo e ricordo sempre che fu in particolare un esponente della Lega, l'onorevole Giorgetti, che diede il contributo più rilevante per l'affermazione di quel principio del pareggio di bilancio. anch'io voterò a favore dello scostamento, ma teniamo presente che non è cambiato, in questo, il mondo: è una situazione che dobbiamo considerare eccezionale. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

su tutte le politiche di bilancio; determina la programmazione economica e finanziaria del nostro Paese; crea le condizioni per dare una prima lettura dell'impostazione della legge di bilancio.

Forse dimentichiamo che per la prima volta da tanti anni stiamo affrontando una programmazione economico-finanziaria senza le clausole di salvaguardia, clausole di salvaguardia, le quali avevano predeterminato danni rilevanti nell'impostazione della legge di bilancio, creando storture e strutture inevitabili per una collocazione rilevantissima di risorse che venivano sottratte alla crescita. Sappiamo bene che questo Governo è nato per impedire l'aumento dell'IVA e per garantire una nuova responsabilità all'Italia anche nella dinamica europea. Credo pertanto che sia evidente a tutti di aggiornamento impatta su due elementi tra di loro differenti. Il primo è una crisi pandemica senza precedenti, che ha determinato un quadro macroeconomico che ha elementi di incertezza rilevantissimi;

esigenze di selezione di misure che fino ad ora non abbiamo mai affrontato. La pandemia, quindi, prima di tutto non meriterebbe una divisione ideologica tra maggioranza e opposizione, né tantomeno un dibattito sempre orientato al passato, secondo il quale c'è un Governo che limita le libertà individuali delle persone. Basta alzare lo sguardo, riguardare il volto di Bergamo, di quando purtroppo eravamo costretti a portare fuori da quella città le bare con i mezzi militari. Sono immagini che non ci consentono contrapposizioni ideologiche senza senso, e lo dico anche all'opposizione. Alziamo insieme lo sguardo, perché di fronte a noi c'è l'interesse generale del Paese; dal modo in cui usciremo dalla pandemia si determinerà il tratto fondamentale del nostro Paese, della sua capacità di dare una risposta a diritti fondamentali molto delicati e importanti (il diritto alla salute, all'istruzione); ne usciremo diversi. Non c'è spazio per una contrapposizione ideologica: c'è bisogno di capire insieme come attraversare la crisi e come dare un volto economico nuovo al nostro Paese. Non possiamo però nemmeno dimenticare che di fronte a noi c'è un'opportunità senza precedenti. Il presidente Monti ha ricordato una fase dell'Europa profondamente diversa rispetto a quella sulla quale stiamo lavorando. Ci sentiamo di poter dire che il Governo italiano e questo Parlamento hanno dato un contributo importante affinché il volto dell'Europa prendesse, all'interno di una pandemia, un indirizzo diametralmente e inversamente proporzionale a un'Europa che ci chiedeva, con il Patto di stabilità, il controllo della spesa. Oggi c'è un Europa che investe, anche attraverso strumenti propri, sul rilancio di un'idea di futuro dell'Unione europea. Io dico, con grande precisione e volontà di essere chiaro su questo punto, il Partito Democratico, proprio nel sostegno a questo Governo, ha nel nuovo europeismo le radici migliori. Oggi è il nostro compleanno, il tredicesimo compleanno del nostro partito. Io credo sia evidente a tutti che, proprio dentro il nuovo europeismo, si fonderà un'idea di futuro importantissima per le generazioni, che guiderà le nuove riforme, a cominciare da quella fiscale. fiscale. Non dobbiamo dimenticare che lo *slogan* dell'abbassamento delle tasse per tutti è, anch'esso, un qualcosa che appartiene al passato. Questa crisi pandemica mostra di fronte a noi esigenze di selettività. Dovremo aiutare settori che rimarranno profondamente indietro, perché le dinamiche della ripartenza saranno diverse. Penso al turismo, penso alle piccole attività commerciali, penso ai servizi. invece, altre dinamiche economiche, a cominciare dalla manifattura, che, sulla dimensione industriale, avranno tassi di crescita differenti. Quindi, dovremo essere selettivi. Affondato il sovranismo, affondata la *flat tax*, affondato lo *slogan* della riduzione delle tasse per tutti, l'intervento che dovremo compiere nella riforma fiscale sarà di riduzione delle tasse sul lavoro, e lo abbiamo fatto. Se renderemo strutturale anche la fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno insieme al cuneo fiscale, già si determinerà una riduzione di pressione fiscale nel 2021. Dobbiamo, però, guardare al più importante investimento per il futuro. Se vogliamo abitare il futuro, oggi è urgente intervenire nella dimensione familiare. Penso all'assegno unico per il figlio. Sono esigenze fondamentali per rimettere in moto le natalità, per dare alle politiche di genere quella trasversalità che meritano, per alzare i livelli di occupazione femminile, per cambiare le caratteristiche fondamentali e i limiti di questo Paese. Le condizioni strutturali che ci hanno impedito di crescere le vogliamo, cioè, rimuovere attraverso la nuova programmazione europea. Questi sono gli elementi fondamentali dai quali noi non possiamo prescindere. Ancora, avremo di fronte a noi una nuova sfida, che non sarà più solo tra Nord e Sud e necessità di recuperare il differenziale, che ovviamente ci porta ad avere un Mezzogiorno che ha bisogno di investimenti infrastrutturali per ridurre le distanze. Questo è vero, sì, ma attenzione, perché di fronte a noi abbiamo le nuove aree interne, che rappresentano le nuove debolezze del nostro sistema territoriale. Per affrontare il tema delle aree interne, che stanno diventando le nuove periferie, dopo la stagione dei tagli lineari e della riduzione della spesa dobbiamo fare un tagliando alla pubblica amministrazione nella sua interezza. Dobbiamo ridare senso alle parole. Autonomia non vuol dire "fai da te". Autonomia significa responsabilità e relazione tra i diversi sistemi territoriali. Se vogliamo rilanciare gli investimenti, dobbiamo definire ambiti ottimali per le stazioni appaltanti e dobbiamo decidere dove assumiamo: non come e quando, ma dove assumiamo per rilanciare gli investimenti. Servono nuove generazioni all'interno della pubblica amministrazione. Serve una sfida espansiva, che abbia, però, al centro, a proposito del diritto fondamentale alla salute, la medicina territoriale. Se vogliamo ridurre le criticità delle aree interne, dobbiamo investire in diritto alla salute nel territorio. Dobbiamo riabituarci, a livello territoriale, a esaminare il bisogno di salute pubblica, che è differente da territorio a territorio. Se non ricostruiamo i distretti socio-sanitari, con una loro autorevolezza e una loro forza, non riusciremo a connettere la responsabilità nazionale del diritto alla salute con le responsabilità gestionali in capo alle Regioni e alle responsabilità in capo ai Comuni e ai territori. Signor Presidente, Presidente, la NADEF che oggi ci apprestiamo ad approvare e il relativo scostamento richiedono una assunzione di responsabilità nazionale. Noi siamo convinti che le politiche adottate da questo Governo hanno dato un primo contributo importante a caratterizzare un nuovo volto dell'Europa. Il modo in cui stiamo attraversando questa pandemia è una distribuzione a pioggia, ma su una visione per aiutare il lavoro, le imprese e le famiglie a costruire un nuovo processo di *green economy*, di digitalizzazione, di futuro del nostro Paese. Se realizzeremo tutto questo, io credo che daremo un grande contributo alle future generazioni e introdurremo finalmente nuove politiche di genere e nuovi investimenti sulle famiglie. E, per poter parlare di futuro, dobbiamo inevitabilmente alzare i tassi di natalità, perché solo alzando i tassi di natalità potremo costruire un futuro migliore per questo Paese. Signor Presidente, signor Vice Ministro, care colleghe e colleghi, innanzitutto la mia solidarietà al Vice Ministro, al Governo, a tutti gli uffici che si occupano del bilancio e ai funzionari del Ministero, perché in sette mesi stiamo approvando uno scostamento di 125 miliardi di euro, che significa più o meno cinque o sei manovre. Rivolgo quindi un plauso comunque per il lavoro svolto fino ad oggi. che qui vicino c'è il teatro Valle, dove, quasi cento anni fa, fu rappresentato per la prima volta un dramma di un grande scrittore italiano: "Sei personaggi in cerca d'autore"

Io credo che abbia detto bene il presidente Monti: e penso che il Parlamento si sia comportato in modo dignitoso. Sono anche contento che molti dei parlamentari seduti qui, che oggi rappresentano o rappresentavano comunque la maggioranza relativa del Paese, abbiano preso coscienza che un conto è star fuori dal palazzo e legittimamente porre dei problemi a chi governa e a chi è nel palazzo, e un conto è poi sedersi e assumersi la responsabilità del governo di un Paese di 60 milioni di abitanti. Non è una metamorfosi quella che avete vissuto: è la presa di coscienza di quanto sia difficile governare e mediare su interessi divergenti. signor Presidente, per quanto riguarda l'opposizione, io penso che in questi sette mesi l'opposizione abbia avuto un atteggiamento quasi sempre costruttivo e leale, ponendo al centro del dibattito politico gli interessi del Paese. Abbiamo votato ben due scostamenti, signor Vice Ministro, con l'impegno - mantenuto in parte o mantenuto per nulla - che il Governo avrebbe aperto un dialogo serio, non con un appello alla responsabilità, perché con la responsabilità non si costruisce un Paese o un progetto politico; con la responsabilità è possibile cavarsela con un voto. Eppure, signor Vice Ministro, non è arrivato nulla. Per l'ennesima volta siamo qui costretti a fare i conti e a chiederci se dobbiamo svolgere un ruolo nella commedia teatrale in cui viviamo: voi portate a noi lo scostamento e noi dobbiamo dibattere se sia il caso di dire al Paese che sono fatti della maggioranza oppure - come io mi auguro per la cultura che mi rappresenta, e ha detto bene la senatrice Conzatti - del popolarismo europeo, se al centro ci devono essere come bussola gli interessi del Paese. Io credo che questo Governo abbia fatto delle cose intelligenti e sagge e delle cose sbagliate. Il ministro Gualtieri l'ha detto anche in televisione, facendo ammenda di alcune negligenze che erano state sottolineate dall'opposizione, in un modo garbato e a bassa voce, come chiedeva il collega dei 5 Stelle. Anche i toni cambiano e questo è importante. Eppure, non c'è stato alcun accoglimento delle nostre preoccupazioni. Guardate che il bazooka dei 400 miliardi non potrà essere attivato; non a caso ne è stato attivato appena il 20 Dicevamo che molte imprese non ce l'avrebbero fatta se non avessero avuto immediata liquidità; e tante stanno chiudendo. Certamente il crollo del PIL del 9 o del 10 per cento è la dimostrazione dell'entità del dramma che stiamo vivendo e non solo della capacità o no di rispondere al dramma che purtroppo che purtroppo stiamo ancora vivendo. Eppure il Governo non ha accolto le nostre preoccupazioni. Noi avevamo parlato di soldi direttamente alle imprese e invece si è dovuta elaborare tutta una strategia che ha comportato per molte aziende la chiusura o il fallimento. Sulla cassa integrazione io non sono uno che finge e si nasconde dietro il dito, perché abbiamo parlato di oltre un miliardo di ore di cassa integrazione in un arco di tempo di due mesi, qualcosa di folle; 11 milioni di italiani l'hanno riscossa, quindi io non ho problemi a dire bravi per certi versi,

Io penso che manchi sempre quel pezzo in più che magari possiamo aggiungere alla dinamica di gestione di questa pandemia.

che si debba chiudere una cerniera e diventare tutti insieme un'unica cosa, ma che in un momento drammatico come questo anche l'opposizione, che rappresenta la maggioranza o la minoranza del Paese (chi se ne importa), possa offrire il suo punto di vista sulla scorta del suo bagaglio formativo, culturale e valoriale. Eppure non lo avete accettato, nonostante molti dell'opposizione abbiano mostrato senso di responsabilità non per far sopravvivere il Governo,

qualunque scellerato sospetto; rivendico in quest'Aula il diritto di chiedere a chi governa e ha la responsabilità del Paese di non trincerarsi ulteriormente. Non credo infatti che la NADEF sia solo un libro dei sogni, però certamente lascia dei punti interrogativi. Fino ad oggi tante delle norme approvate, come si suol dire, non sono atterrate per le difficoltà burocratiche. Come pensate di superarle, soprattutto oggi che non avete la maggioranza del governo dei territori?

oggi non c'è. Non c'è quella cultura politica che permetta di poter dire a due terzi del Parlamento che stiamo condividendo un percorso comune in un momento drammatico, con il rischio che vi sia un ritorno della pandemia,

per poter gestire e governare un territorio, ma lo si fa perché c'è un'emergenza sanitaria che in questo momento è prevalente rispetto alle libertà individuali. Io sono al di fuori di queste polemiche e mi sento anche un po' un pesce fuor d'acqua, però date almeno ragione a chi vi chiede questo, perché se non lo farete è ovvio che tutti quanti continueremo a commettere un errore per il Paese. Qui stiamo indebitando per 120 miliardi le future generazioni, i nostri figli, e come pensate di farlo da soli,

Con tonalità diverse, noi stiamo chiedendo questo, niente di più, signor Presidente. Io mi auguro che il disegno di legge di bilancio che arriverà nei prossimi giorni sia un'occasione per aprire un tavolo serio nell'interesse del Paese, non della sopravvivenza di questo Governo.

le linee guida per il Piano nazionale di ripresa e resilienza; oggi, di fatto, dobbiamo aggiustare il tiro perché le previsioni fatte non erano corrette; e domani ci troveremo a discutere della legge di delegazione europea. Si tratta, da punti di vista differenti, di tre passaggi fondamentali in vista della prossima legge di bilancio. quello che è evidente è che c'è sì la stessa narrazione da parte del Governo e della maggioranza, ma senza che ci sia un filo conduttore e un progetto coerente e complessivo. Questo è quello che da giorni in Commissione, in Aula e in tutte le occasioni stiamo cercando di sottolineare: lo sta facendo la Lega così come lo stanno facendo le altre forze di centrodestra.

tranquilla apprensione o, per dirla in termini politici più consoni ai *social network*, potremmo dire che l'*hashtag* è: «italiano stai sereno». *(Applausi)*.

ci ha sottolineato - non me ne voglia per la battuta - che avrebbe tralasciato numeri e percentuali per concentrarsi sugli aspetti fattuali. Questo è bene, tuttavia - permettetemi - con una battuta si potrebbe dire che il confine fra fornire dati e dare i numeri - perché questo sta facendo la maggioranza in Aula - è molto sottile. Quello che dovremmo dire è che oggi non abbiamo certezze; ci sono delle contraddizioni - e che fra poco dirò - anche nella

i tempi e i costi - perché dei costi ci saranno per il Paese - delle risorse che saranno messe in campo. La Nota di aggiornamento dovrebbe riguardare scenari e prospettive ed analizzare le misure adottate. Quanto noi dobbiamo fare un'operazione verità; l'ha fatta in parte il vice ministro Misiani poco fa in Commissione bilancio. La verità è che, a prescindere dall'emergenza sanitaria e dalla crisi economica scaturita, la la situazione italiana era già critica e c'era già una bocciatura sostanziale delle politiche avviate da questo Governo. Tanto è vero - diceva il Vice Ministro - che l'obiettivo non è semplicemente quello di tornare al livello *pre* crisi, ma uscire da una stagnazione lunga vent'anni che l'Italia deve sconfiggere e superare. Sull'obiettivo nulla da ridire, però sicuramente lo scenario che viene tracciato non è esattamente coerente con tale obiettivo. Leggo dalla relazione. La relazione già oggi prende atto di un peggioramento rispetto alla previsione di aprile e dice che la ripresa economica è più contenuta rispetto a quanto previsto dal DEF e porta a una riduzione del PIL reale nel 2020

il problema che ha portato a questa previsione? Si dice «Il principale motivo della previsione al ribasso per il 2020 risiede nella contrazione più accentuata del PIL nel secondo trimestre, conseguente alla durata del periodo di parziale chiusura delle attività produttive in Italia e alla diffusione dell'epidemia su scala globale superiori la previsione. Tuttavia, nella relazione si intravede un cauto ottimismo poiché dice che la nuova previsione sconta inoltre i progressi del contrasto dell'epidemia, l'ipotesi di una gestione controllata dei focolai che consentirà di non arrivare a un *lockdown* a livello nazionale, l'arrivo di vaccini anti-Covid entro il primo trimestre 2021 e una loro distribuzione su larga scala. Ma questa previsione è largamente irrealistica. di ieri la notizia della sospensione da parte di alcune case farmaceutiche addirittura della sperimentazione sui vaccini. Dire oggi che si fa una previsione quasi quasi positiva, o meno negativa, perché si dà per scontato l'arrivo di un vaccino nel primo trimestre e la sua diffusione su larga scala è irrealistico. Questa è una delle condizioni di scenario che sconta una previsione che, a nostro giudizio, rimane, purtroppo, ahimè, eccessivamente ottimistica. C'è un altro passaggio sul quale vorrei soffermarmi. Qual in termini logici - quasi da sillogismo aristotelico - il punto di partenza del Governo? Abbiamo dato stimoli, gli stimoli funzionano; torneremo a crescere. Bene, queste premesse alla base del ragionamento non sono non sono corrette. Perché? Intanto gli stimoli che abbiamo dato, di fatto, a oggi, sono interventi di sostegno, interventi assistenziali piuttosto che vere e proprie iniezioni di investimenti che possano rivedere la situazione. D'altro canto, il fatto che stiano funzionando è tutto da dimostrare. Questa contraddizione è talmente evidente che, persino nella relazione, a pagina 2 si dice una cosa, e a pagina 5 se ne dice un'altra o si lascia intendere l'esatto contrario. Ce lo dite, allora, se nel fare riferimento alla previsione avete tenuto conto o meno degli investimenti a livello europeo? A pagina 2 si dice che la programmazione finanziaria tiene altresì conto degli interventi straordinari per il sostegno e il rilancio dell'economia che il Governo intende concordare con la Commissione europea attraverso la presentazione a ottobre dello schema di Piano Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito delle procedure per l'accesso ai fondi stanziati con il programma *Next generetion EU,* dotato di 750 miliardi; dall'altra parte, si dice esattamente il contrario, giocando sulle parole, basandosi su quel filo sottile a cui facevo riferimento all'inizio,

Tiene conto o meno dell'impatto che avranno le risorse europee e che saranno utilizzate? Alla fine, il fulcro della previsione fondamentale sarà il rapporto *deficit*-PIL nel 2021, perché è evidente che per riavere la crescita, in un momento di stagnazione della domanda privata, dovremo puntare sugli investimenti e sul ruolo del pubblico, e ci mancherebbe altro, ma quale sarà l'effetto moltiplicatore? In sintesi, per ogni euro di *deficit* in più, quale sarà la crescita del PIL attesa? Sarà inferiore o superiore a 1? Quell'1,3 previsto tiene conto solo delle risorse nazionali o anche di quelle europee, che di fatto sono una esternalizzazione del costo? Ce lo dite come stanno veramente le cose da questo punto di vista? A noi non interessa discutere sulla previsione dell'entità del disastro: ripeto, restare sopra o sotto il 10 per cento di calo del PIL non credo sia ciò che interessa agli italiani che devono mettere insieme il pranzo con la cena, che hanno problemi a intravedere un futuro per i propri figli o, per chi deve tirar su la serranda e resistere a una crisi economica devastante. Quello che ci interessa - dicevo - è lavorare per evitarlo, il disastro: esattamente quello che il Governo non ha fatto fino adesso e si ostina a non fare andando avanti da solo, senza il minimo coinvolgimento delle opposizioni e del Paese.

il nostro Paese, o meglio il mondo intero è stato travolto dal Covid, una pandemia che ha spezzato la società, gli affetti, il modo di vivere e di pensare, l'economia, il commercio, la mobilità internazionale. Lo scenario macroeconomico internazionale, illustrato nella Nota, evidenzia che nella prima metà del 2020 l'economia mondiale ha subito, a causa del Covid, la battuta d'arresto più profonda dalla Seconda guerra mondiale, conseguente al blocco delle attività economiche. Nonostante gli interventi straordinari messi in campo dai Governi e le misure di politica monetaria introdotte dalle Banche centrali, il blocco produttivo ha determinato una contrazione del PIL e del commercio mondiale, rispettivamente del 3,5 per cento e del 2,7 per cento nel primo trimestre dell'anno, rispetto al trimestre precedente. Tale contrazione si è andata accentuando nel secondo trimestre, con un calo del 5 per cento del PIL e del 12,5 per cento del commercio mondiale. La caduta del PIL ha interessato tutte le principali economie avanzate, come gli Stati Uniti e il Giappone,

che avendo riattivato l'economia già all'inizio di aprile, ha registrato una crescita del 3,2 per cento, su base tendenziale, nel secondo trimestre. Una graduale ripresa, più sostenuta delle attese, si è registrata a partire dai mesi di maggio e giugno, col riavvio delle attività produttive, ma con un andamento disomogeneo tra i vari Paesi.

Purtroppo il livello del PIL, in termini reali, potrebbe rimanere inferiore del 3,5 per cento rispetto a quello atteso nelle proiezioni di dicembre. Secondo i dati riportati dalla Nota, gli indicatori disponibili registrano un andamento in crescita nei mesi estivi dell'indice della produzione industriale, con un anche nel settore delle costruzioni, con un aumento del 3,5 per cento. La questione è se, nel futuro prossimo, nel Paese perdureranno le disuguaglianze, tra Nord e Sud, tra ricchi e poveri, tra chi ha accesso al futuro digitale e chi no, così come ci ha indicato per una volta l'Unione europea. La pandemia ha rimescolato le carte e ha rimesso tutto in gioco. Qualche mese fa, tutte le previsioni interne e internazionali dicevano che avremmo avuto un grande tonfo, ma altri Paesi, come Francia e Spagna, stanno peggio di noi. Le rigide regole di controllo del virus fissate dal Governo e il comportamento virtuoso dei nostri cittadini ci stanno forse mettendo al riparo da un nuovo *lockdown*, quasi certo in Spagna, Francia, Belgio, Regno Unito, Ungheria e Repubblica Ceca, probabile in Germania. In contemporanea, le risorse messe in campo per sostenere l'economia e soprattutto per impedire l'allargamento delle forbici sociali, probabilmente riusciranno a non far crollare del tutto la domanda interna, principale volano per la ripresa economica, come la soppressione delle clausole salvaguardia, l'esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019, del primo acconto IRAP 2020, le agevolazioni per interventi di efficientamento energetico, i benefici fiscali per l'acquisizione di servizi turistico-ricettivi da parte delle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro, gli sgravi contributivi volti a sostenere il livello occupazionale, il superbonus. La manovra prevede significativa risorse per il sostegno dell'occupazione e dei redditi, il completamento del finanziamento del cuneo fiscale, il rifinanziamento del taglio contributivo al Sud, il rifinanziamento delle cosiddette politiche invariate, mentre ci sono componenti importanti della programmazione, come l'introduzione della riforma fiscale. A proposito di Europa, finalmente possiamo dire che le linee guida provenienti da Bruxelles non sono sulla falsariga della religione neoliberista e questo lo si deve anche al Governo e alla maggioranza. *(Applausi)*. Questo è un grande successo che può vantare l'Italia, come ci ha riconosciuto anche l'Organizzazione mondiale della sanità, per aver per aver combattuto questa pandemia. La "zattera Italia" è stata trascinata per tre decenni dalla corrente impetuosa del neoliberismo, grazie anche alle vele forniteci dall'Europa, verso il baratro dell'autodistruzione. Il Covid ci ha mostrato tutto ciò e ci ha fatto finalmente aprire gli occhi. È arrivato il tempo di andare controcorrente e di cambiare le vele. È stata l'Europa a fornircele: bisogna cambiare paradigma. Ieri, signor Presidente, lo *spread* è sceso a 120, con rendimenti triennali a meno 0,14: una sorta di nemesi per i piazzisti del MES, quel feticcio agitato a meri fini di propaganda che nessun Paese UE ha richiesto. *(Applausi)*. Ringrazio di cuore il ministro Gualtieri per la saggezza dimostrata dopo aver compreso che questo *totem*, evocato come la panacea di tutte le questioni sanitarie proprio da parte degli "Attila" del sistema sanitario, è antieconomico, se non una vera e propria sciagura per l'Italia. Sul MES non c'è bisogno di qualche bocconiano per smentirne la convenienza economica con gli attuali tassi; basta un semplice pallottoliere, quell'abaco antico utilizzato per i calcoli fin dal ventunesimo secolo avanti Cristo. Bisogna cambiare paradigma: non può essere la finanza a dettare l'agenda alla politica e ai Governi democratici. Ieri in Commissione bilancio è stato presentato un documento dal direttore generale del Tesoro, dottor Rivera, sulla genesi degli strumenti derivati. una tabella che rappresenta la plastica subalternità della politica e dei Governi alla finanza e all'oligarchia dei banchieri. Dal 2011 al 2019, mentre alcuni Paesi hanno guadagnato dai contratti derivati quasi 20 miliardi), l'Italia, grazie a contratti capestro, ha pagato alle banche di affari 45 miliardi di euro. Ripeto: 45 miliardi di euro, con direttori generali e ministri dell'economia poi assoldati dalle banche di affari, da Mario Draghi a Vittorio Grilli e a Domenico Siniscalco. Cari colleghi, credo che debbano essere raccolte le richieste di azioni comuni per fronteggiare la pandemia del presidente Schifani e del senatore Salvini, a patto che finiscano gli insulti, la denigrazione, la mistificazione sull'operato del Governo, così come avvenne nel secondo dopoguerra per scrivere la Costituzione, quando Nenni, De Gasperi e Togliatti, non rinnegando le rispettive ideologie, trovarono un compromesso nella Costituente, rammentando che quei *leader* non ricorrevano all'insulto, ma al rispetto reciproco. reciproco. Ora come allora, per superare una sciagura planetaria analoga ad un conflitto mondiale che ha colpito l'economia di tutto il mondo, abbiamo, specie in Italia, l'occasione storica per riscrivere gli assetti delle due Camere, per cento dei «sì» al *referendum* costituzionale sul taglio di deputati e senatori, i Regolamenti parlamentari e la legge elettorale, che non devono essere come in passato appannaggio della maggioranza, ma patrimonio comune. In quest'epoca immorale delle disuguaglianze sociali, dove la pandemia ha messo in crisi un modello neoliberista, in questa Italia disuguale occorre restituire fiducia,

in occasione di un viaggio in Europa, rimasi colpito da una frase di un girovago, un saltimbanco che incontrai a Marsiglia ad uno spettacolo teatrale: *Je ne travaille pas pour l'argent, je travaille pour l'amour* (tradotto: non lavoro per il denaro, lavoro per amore). Ecco, in quest'epoca di avidità *(applausi)...*arrivismo, mistificazione, sopraffazione, distruzione dei valori fondanti di una società, nell'era del neoliberismo e del globalismo che hanno messo in soffitta i tre sacri principi dell'illuminismo, base delle Costituzioni democratiche, quali libertà, uguaglianza e fraternità, con il primato dell'uguaglianza, perché senza di essa non ci sono né libertà ne fraternità, nell'epoca della spietata lotta per il potere il potere che genera odio sociale, globalizzazione dei capitali che ha creato la globalizzazione della povertà, noi del MoVimento 5 Stelle lavoriamo spinti dall'amore verso l'Italia ed il popolo italiano, coltivando quei valori di uguaglianza, solidarietà e rispetto reciproco. *(Applausi)*. Mi permetto di rinnovare un appello alle opposizioni democratiche per lavorare insieme, per perseguire gli interessi generali ed il bene comune dell'Italia, ricostruendo dalle macerie, come i nostri padri nel dopoguerra. Grazie dell'attenzione.

senatori saggi e autorevoli, che mi hanno consentito anche di orientare quello che dirò adesso. Non mi ricordo se in quest'Aula è stato commemorato Emanuele Severino, quando purtroppo è stato richiamato dal Signore; se fosse presente, di sicuro mi aiuterebbe a dire quello che proverò a dire. La realtà di questo pianeta è fatta di due consistenze: da una parte c'è la natura e io, da credente, dico che la natura è tutto ciò che Dio ci ha messo; dall'altra parte c'è la civiltà, la cultura o la tecnica ed è tutto quello che l'uomo aggiunge. Noi abbiamo patito la rivoluzione della natura. La pandemia, nei fatti, è un ribellarsi della natura, che ha determinato una rottura della civiltà. L'ordinamento, la politica, la legislazione devono essere capaci di trovare soluzione rispetto alla rottura di civiltà. Cosa si è determinato? Abbiamo messo in campo misure straordinarie, riportate anche nella fotografia della Nota ma siamo davanti ad un'altra difficoltà: se la NADEF è una fotografia, così come la legislazione prevede, noi siamo in una condizione nella quale la fotografia non ce la fa più a contenere, a rilevare la realtà. Vi sarebbe bisogno di una specie di ripresa cinematografica per la velocità dei cambiamenti. Tutto quello che è stato condiviso tre mesi fa rischia, dopo novanta giorni, di non resistere più. Quali sono i numeri riportati in questo documento? Noi sappiamo che alcune misure normative hanno determinato un recupero di liquidità a favore di imprese e famiglie; numeri straordinari, mai concepibili prima. Abbiamo determinato più volte lo scostamento della consistenza di bilancio e lo faremo di nuovo anche in questa circostanza; abbiamo prefigurato che il recupero della normalità pre Covid-19 circa il PIL, che è l'insieme dei beni e dei servizi prodotti da un Paese, avverrà avverrà soltanto nel 2023. È questo ciò che dimostrano le prefigurazioni. La NADEF è, nei fatti, uno sforzo di programmazione, che però è caratterizzato, in questa fase, da oggettiva debolezza: non sappiamo come evolverà la capacità distruttiva di questo contagio da Covid-19. Io sono europeista, il che vuol dire che sono "anticonfinista". L'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che è competenza dell'Europa prevenire e reagire rispetto a flagelli e a pandemie.

non gli Stati membri nazionali. C'è un cammino su questo fronte, che ha visto protagonista l'Italia: la grande consistenza di copertura del *recovery plan* è un obiettivo conseguito rispetto a questa nuova idea dell'Europa,

un luogo in cui si parla, cioè un parlatoio, ma un Parlamento, in cui si compongono i punti di vista dialettici, per collocare in alto la linea della virtù che poi produce la norma. la norma. In allegato alla NADEF abbiamo una serie di obiettivi normativi. Ne cito tre di mio grande interesse anche per il ruolo che ho nella Commissione finanze. finanze. Nel corso dell'esercizio parlamentare che si inaugurerà a gennaio avremo l'aspettativa di una legge delega riguardante la riforma fiscale e tributaria. Voglio dire a chiare lettere, riportando le parole di autorevoli intellettuali del diritto, che la legge delega è l'unico strumento per affrontare la complessità di una riforma fiscale. L'alternativa è è ciò che abbiamo già conosciuto come prodotto normativo (il decreto-legge, che costringe quasi faccia al muro il lavoro parlamentare) o la normalità del lavoro parlamentare che non ce la fa ad arrivare alle altezze della *téchnè* che richiede un processo di riforma fiscale e tributaria. Lo stesso dicasi per la legge la legge delega riferita alla riforma della giustizia tributaria, che da più parti molti ci chiedono. In terzo luogo, sono molto interessato rispetto a quanto scritto nella NADEF che il 2021 sarà l'anno nel quale metteremo a segno un'agenda per la semplificazione, che è la parte corposa riferita alla legge sulle semplificazioni. Noi manchiamo di 500.000 risorse umane; abbiamo in pancia 130 miliardi di euro prima del *recovery fund*.Con le risorse del *recovery plan* arriveremo a circa 300 miliardi di euro per spingere la ruota dell'economia. Se non c'è la funzione amministrativa, non ce la faremo ed è bene allora che sia scritto nel documento che ci occuperemo anche dell'agenda delle semplificazioni. Per queste ragioni parlo a favore, sapendo che l'Italia ha vissuto tre momenti di rottura di civiltà. Il primo è stato appena dopo la Seconda guerra mondiale nel luogo che diede anche origine alla Costituente, che era la parte duale che metteva insieme tutte le appartenenze partitiche per dare luogo al prodotto straordinario che è stata la Carta costituzionale. la lotta del sistema Paese rispetto al fenomeno violento del terrorismo. Anche allora ci fu uno sforzo straordinario di convergenza, prendendo atto del rischio, della rottura e della paura che c'era nel Paese. Questa è la terza volta e la terza fase. Cosa deve accadere affinché ci sia un allineamento verso l'alto dei punti di vista politici di tutti? Io mi aspetto che, a partire dalla NADEF e dal bilancio che dovremo anche mettere in cammino per il 2021, ci sia uno sforzo di convergenza di tutti

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza del 2020 la riteniamo anche noi plausibile sulla base delle tendenze attuali, a meno di un ritorno del *lockdown*. Nelle aziende, quando si preparano i *business plan*,

e c'è il *worst case*, ovvero cosa accade se la situazione si mantiene tale o addirittura peggiora. Secondo me, questo aspetto manca, proprio perché siamo in una situazione emergenziale

Vogliamo parlare del settore del turismo, della ristorazione, dei servizi, di tutto il mondo del lavoro a tempo determinato che è sparito? alle situazioni di crediti messi a disposizione delle aziende, finanziamenti, ma sempre debiti sono, che esse non vanno a «tirare» perché sempre di debito si tratta.

Mi dispiace che non ci sia il professor Monti, ma vedo il collega Lannutti che l'ha richiamato. Anche ieri il senatore Renzi

dell'intolleranza e di tutto e di là ci sia il saggio, il buono e il bello. No, io questo lo rifiuto categoricamente. In questo momento, proprio perché siamo in emergenza, c'è bisogno di tutti. c'è bisogno di tutti. C'è bisogno dell'apporto serio, responsabile, ragionato e profondo di tutti. Noi, come di Forza Italia siamo inseriti nell'ambito del filone del Partito popolare europeo.

che ha richiamato la sua esperienza di Governo; abbiamo appoggiato anche noi quella fase storica, ma qualcosa non ha funzionato se i risultati, col senno di poi, sono quelli che abbiamo visto pre- Covid. Cosa non ha funzionato? Non ha funzionato, secondo il mio modesto parere, il fatto che la carenza di politica, quella con la P maiuscola, che caratterizzava quel Governo, l'aveva reso debole; l'aveva reso gradito agli occhi della tecnocrazia europea, ma non era permeato nel substrato della nostra Nazione *(Applausi)*, che è una realtà eterogenea e complessa che deve considerare vari interessi e varie realtà. Mi accingo ora ad alcune considerazioni nel merito. Abbiamo fatto tutta una serie di decreti, che avete ricordato tutti. con grandi annunci; tutte le sere il presidente Conte ci intratteneva con le sue conferenze stampa, con tutti i favori delle telecamere nazionali e locali. Oggi «Il Messaggero» riporta quanti decreti attuativi mancano per dar voce, sostanza e concretezza a quelle norme che rimangono edittali. Signor Vice Ministro, ne cito due, molto banali.

Ripeto, sono 380 i decreti attuativi che mancano. Gira la voce - ma non abbiamo la forza di dirlo

che non riusciremo a tradurli in atti concreti. Signor vice ministro Misiani, signor Sottosegretario, non si potevano bloccare le tariffe per l'energia elettrica e il gas in questo periodo di recessione, in cui le famiglie sono in grossissime difficoltà?

è il Governo che deve dare l'*input* e dirigere questo passaggio, affinché la macchina faccia un superlavoro.

questo è il problema: bisogna agire subito. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa: si chiede alla pubblica amministrazione di dare qualcosa in più.

completamente cambiata; lo chiediamo ai bambini e ai ragazzi che sono nelle scuole; lo stiamo chiedendo a tutti. Lo possiamo chiedere anche ai Ministeri? Ci sono tutte le intelligenze e le capacità, bisogna che facciano un superlavoro, perché l'Italia ne ha bisogno.

tutti siamo pronti a fare la nostra parte. In Commissione sono stata bacchettata, perché mi sono permessa di dire che, a mio avviso, bisogna anche curare

aumentano e che si fanno moltissimi più tamponi, quindi i casi positivi sono molti di più; ma bisogna distinguere quali sono i casi positivi asintomatici da quelli sintomatici, perché il costo di tutte le misure dipenderà anche da questo

10-12 esperti tutti i giorni, di cui uno dice una cosa, uno l'esatto contrario: la gente normale, che non è laureata in medicina o che non vuole approfondire, come fa a orientarsi? È disorientata, è impaurita.

Questo equilibrio è assolutamente necessario, perché da tale percezione dipendono anche i comportamenti delle persone e le propensioni al consumo. Sono stati dati grandi aiuti, ad alcuni addirittura per la sopravvivenza, ad altri perché potessero comunque non solo vivere con un minimo di tranquillità, ma anche sostenere la domanda interna; se c'è però questo terrore, ciò incide non solo sulla depressione delle persone, ma addirittura sull'economia, perché sappiamo benissimo che le aspettative delle persone sono una variabile che entra nell'economia, a volte anche pesantemente.

Il viceministro Misiani, su alcuni, ha detto: effettivamente qui non ce l'abbiamo fatta, ma dovremo pensarci in legge di bilancio. Per me, questo

i suggerimenti dell'opposizione e che bisogna avere il dialogo: questo avviene se ci si parla e ci si ascolta. Ieri Matteo Salvini lo ha ribadito. Noi ci siamo, con responsabilità, come sempre. Lo abbiamo dimostrato, nonostante l'andamento talvolta

di voci di territori e di problematiche magari più di altri, quindi questo confronto dev'esserci. Dipende però da voi far diventare tale passaggio un momento importante per questa Istituzione.

rendere necessaria questa unione di intenti, non solo per il breve termine. Adesso stiamo pensando di adottare provvedimenti tutti insieme per arginare un'eventuale seconda ondata ma, allo stesso tempo, dobbiamo essere tutti così lungimiranti da pensare a quello che sarà il Paese dopo. Dobbiamo cioè permettere, ad esempio, alle piccole e medie imprese, visto che il nostro tessuto è fatto da questi soggetti, di essere così resilienti da poter ripartire, appena sarà possibile, con una quasi normalità, perché così lo si potrà fare. Ci sono aziende, per loro fortuna, così *smart*, così avanti e così strutturate che

però, sono ancora indietro. Non possiamo guardare solo il presente, dimenticando l'obiettivo di lunga durata; dobbiamo programmare quello, per la scuola, per l'edilizia, per il lavoro dei giovani e per tutte queste categorie fondamentali. Se, finita la pandemia, saremo soltanto disorientati, allora sarà davvero la fine. Spero che la pandemia

pur non avendo vissuto la stessa drammaticità delle zone di Bergamo, di Cremona e delle aree più colpite. Spero che ci sia tanta responsabilità da parte di tutti e che non si senta mai più, da nessuna parte,

l'ospedale Fiera Milano anche ad altre Regioni. Penso che questo sia l'atteggiamento giusto, di chi supera le cattiverie e le meschinità e pensa al bene delle persone italiane, di qualunque parte siano. Prendiamo esempio dalla Lombardia.

un collega di opposizione ha ricordato a tutti noi, anche a proposito della NADEF, che nessuno avrebbe mai immaginato di aver timore dell'altro e di andare a cena con gli amici o di parlare con la mascherina;

Mi rivolgo soprattutto all'opposizione: dove si può agire la responsabilità meglio che in una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 in un tempo eccezionale? Sono stati citati molti nostri Padri costituenti: De Gasperi, Togliatti, Nenni; sarebbero però da citare anche grandi donne, grandi nostre madri: Tina Anselmi, Nilde Iotti, Giglia Tedesco. Giglia Tedesco. *(Applausi)*. Questi grandi uomini e queste grandi donne non sono nati Togliatti, Nenni, De Gasperi, Iotti, Anselmi e Tedesco, ma lo sono diventati per la loro responsabilità nell'agire.

A questo proposito, l'Italia, come si ricorda nella NADEF, deve tener conto della raccomandazione n. 1 del Consiglio dell'Unione europea del 20 luglio 2020: rafforzare la capacità e la resilienza del Sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture. Il nostro Paese deve colmare, sì, la carenza di investimenti pubblici nell'assistenza; l'assunzione del personale sanitario, in rapporto alla proiezione occupazionale in questo settore, deve superare l'imbuto formativo dei medici specializzandi. La terribile epidemia - lo diciamo, ma dobbiamo agire anche questo - deve essere per noi un'opportunità.

(penso al Sud). Ho ricevuto l'altro ieri una delegazione di sindaci dell'entroterra cosentino, che hanno rappresentato il loro grido di dolore (si sono espressi con queste parole) paura della mancata assistenza ai loro concittadini. Dobbiamo rovesciare le politiche sanitarie, mettendo al primo posto la prevenzione primaria, la medicina di territorio, la digitalizzazione, i servizi domiciliari. Dobbiamo dare il massimo sviluppo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la NADEF richiama il disegno di legge collegato alla legge di bilancio su questo tema. Dobbiamo avere un piano generale dei trasporti pubblici: questo Governo dovrà farlo molto bene nella legge di bilancio, perché sappiamo che molti contagi avvengono durante il trasporto.

alla salute e allo sviluppo. C'è poi la ricerca. Come diceva molto bene ieri la senatrice Cattaneo in Aula, un Paese che non investe in ricerca non ha futuro; questo nella legge di bilancio dobbiamo affrontarlo in maniera molto forte. Dovremo pensare anche a forme di partecipazione dello Stato come socio garante per quelle realtà sono convinta che avremo più posti di lavoro in alcuni settori, ad esempio nel farmaceutico, nella ricerca, nelle imprese di sanificazione, nel digitale. una politica occupazionale strettamente connessa a una industriale di investimento in questi settori. La senatrice Conzatti stamattina diceva di andare oltre alla NADEF e alla alla legge di bilancio; anche il senatore Renzi ieri affermava che affronteremo questa difficoltà, soprattutto anche occupazionale, che riguarderà il lavoro dei nostri giovani, se avremo una prospettiva.

disagio nella propria vita esistenziale sa che soltanto costruendo una prospettiva può uscire da una condizione di difficoltà che la NADEF e la legge di bilancio avranno questa prospettiva, rivolgo un appello al Governo e ai miei colleghi di maggioranza per dire che dovremo avere un atteggiamento più accogliente nei confronti delle istanze dell'opposizione, così usciremo tutti insieme da questa crisi che riguarda la nostra umanità, perché ci formiamo in relazione con l'altro.

cita la misura dell'assegno unico universale per i figli nell'ambito di uno degli interventi più articolati, ovvero la riforma fiscale. Non entro nel merito della programmazione generale della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, ma mi concentro sulla misura, a lungo attesa, dell'assegno universale per i figli. Facciamo un passo indietro per contestualizzare il tutto. Il 20 luglio scorso è stata approvata all'unanimità

Anche Fratelli d'Italia ha espresso il suo voto favorevole alla Camera sulla misura dell'assegno unico. Lo ha fatto per sostenere le famiglie e favorire la natalità, come abbiamo sempre fatto con le nostre proposte di legge e con tutti i nostri emendamenti ad ogni disegno di legge del Governo e ai disegni di legge di bilancio. Devo anche ribadire che avremmo preferito una norma immediatamente operativa e non i tempi incerti e lunghi di un disegno di legge di delega. La criticità dei tempi lunghi, inoltre, non riguarda solo la misura dell'assegno, ma tutto il pacchetto del *family act*, perché, per esercitare la delega, l'Esecutivo si è preso praticamente due anni di tempo e quindi al momento il tutto ci appare - lo dico con paura - come una scatola vuota. Desidero inoltre introdurre un'altra considerazione tecnica. Stiamo assistendo ad un abuso dei decreti-legge; vi si fa un ricorso eccessivo, direi compulsivo, ma purtroppo si moltiplicano anche i ricorsi, come nel caso di specie, ai disegni di legge di delega, con i quali le Camere delegano il Governo a legiferare in determinate materie. Insomma, si tratta di uno strumento che sposta il baricentro della produzione legislativa dal dal Parlamento all'Esecutivo: una sventagliata di disegni di legge di delega con la quale il Governo prima ipoteca l'attività legislativa, relegando il Parlamento a un ruolo sempre più marginale, e e poi la svolge in parte. Queste che ho letto non sono parole mie, ma un'annotazione comparsa sul «Corriere della Sera» l'8 ottobre scorso in un interessante commento a firma di Enrico Marro.

deleghe dell'elenco attuale provengono dalla lista dell'anno scorso e tra quelle inevase e rimaste sulla carta c'è proprio quella cruciale della riforma fiscale, cui si coordina l'introduzione dell'assegno universale. Torniamo a quella paura della scatola vuota a cui facevo riferimento all'inizio. Al momento, signor Ministro, sulla misura non sono previste coperture economiche e sono vaghe le indicazioni sull'importo minimo garantito al mese per ogni figlio. Quindi è necessario individuare le risorse necessarie nella prossima legge di bilancio, alla luce anche dei decreti attuativi, nonché - come detto - il si accompagni ai tempi della riforma fiscale. Domanda: qual è la *roadmap* che l'Esecutivo ha individuato perché si passi dalle parole ai fatti e affinché l'assegno unico diventi una realtà e raggiunga materialmente le famiglie? Insomma, l'eterno tema:

tempi e cifre in senso reale. Come dicevo, è una misura molto attesa da un Paese, l'Italia, che nelle statistiche di aspettativa di fecondità vorrebbe fare figli, ma poi rinuncia a farli, e non per edonismo o per egoismo, ma perché sono un costo economico, che direi diventando sociale ed esistenziale. Credo che sia necessario concentrarsi su tale questione, considerato che l'Istat ci ha ricordato che nel 2019 abbiamo raggiunto il *record* negativo dal punto di vista demografico, con un calo del 4,5

è quello di non discriminare coloro che oggi non riceveranno nulla nel prossimo assegno. Soprattutto, è stata calcolata la necessità di uno stanziamento aggiuntivo di 6 miliardi. Questo è il punto: dove si prenderanno? Qualche maligno dice dice che il Governo dovrà scegliere se darli al Sud con il taglio del cuneo fiscale (che dev'essere confermato dall'Unione europea) o alle famiglie per fare figli. Mi auguro che il Governo non si trovi a dover fare questa scelta. Signor Presidente, il punto il punto è la visione. Anche nel *recovery fund* le politiche sociali e familiari sono centrali o sono cenerentole? Fratelli d'Italia ha chiesto che siano centrali e che ci sia un'attenzione speciale nell'ambito degli oltre 200 miliardi che l'Italia dovrà spendere per resilienza e ripartenza. Infine, la volontà e la determinazione dell'Esecutivo ci sono o per investire sulle famiglie e sulla natalità, per invertire la rotta demografica e quel *record* negativo, insomma per sostenerle davvero? Concludo, senza polemica, su questo tema: c'è la paura che i fondi per questa misura dell'assegno unico non arrivino e non ci siano, né si trovino i 6 miliardi aggiuntivi necessari. La paura - che per noi è, anzi, una convinzione - è che non abbiate capito che serve un piano di salvataggio della famiglia e della natalità; non lo capirete, se non avrete una visione di sistema, con politiche organiche di sostegno alla famiglia e alla natalità.

Signor Presidente, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza che stiamo per votare ci presenta un quadro di politica fiscale che si mantiene - e non potrebbe essere altrimenti - fortemente espansiva. Questo avviene anzitutto con un ulteriore scostamento dal rientro verso l'obiettivo di medio termine; scostamento che - è giusto ricordarlo - è perfettamente in linea con la clausola di salvaguardia generale del Patto europeo di stabilità e crescita che l'Unione europea ha deciso giustamente di estendere, anche perché, a differenza di altre crisi, c'è la consapevolezza a livello europeo che gli Stati nazionali devono essere lasciati in grado di mantenere politiche espansive per uscire dalla crisi. Vi sono, poi, le risorse del Next generation EU, che la Nota di aggiornamento considera e i cui effetti comincia a stimare; anzi, con un effetto di moltiplicatore fiscale sulla crescita del Paese

è anche utile che la politica abbia consapevolezza che, dall'utilizzo di questi fondi, dobbiamo essere in grado di attivare un moltiplicatore fiscale ben maggiore, se vogliamo rimettere il Paese su un sentiero di crescita. Da qui viene il primo elemento politico di questa discussione sulla Nota di aggiornamento, secondo me, ovvero che i soldi dello scostamento, i soldi europei, non vengono da Marte; vengono dal futuro, perché li stiamo chiedendo in prestito alle future generazioni di europei e di italiani. Neanche i sussidi a fondo perduto vengono da Marte, come pure i trasferimenti dell'Europa, che giustamente rivendichiamo come Paese ad alto debito, perché abbiamo bisogno di quelle risorse, che non impattano sulla sostenibilità del debito e sono una risposta giusta e forte dell'Europa (un embrione di unione fiscale che completa quella monetaria,

Dobbiamo quindi sentire il peso della responsabilità di spenderli bene, mettendo al centro i giovani di oggi e le future generazioni, da cui questi soldi arrivano. Questo elemento ha un'implicazione: dobbiamo velocemente cambiare passo, non perché il primo non fosse giusto e necessario, ma perché adesso ne serve uno diverso. Da una logica emergenziale, che giustamente mirava a risarcire persone e le imprese più colpite da una crisi terribile, come quella che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, dobbiamo passare a una progettuale, che metta al centro una visione di crescita del Paese. Certo, dobbiamo farlo con serietà e gradualità, come ci invita a fare anche la Nota di aggiornamento nel quadro di finanza pubblica. Gradualità vuol dire che adesso dobbiamo mettere al centro tre ingredienti: il primo è una serie di interventi ancora emergenziali, ma selettivi, rispetto ai settori più colpiti (turismo, spettacolo e una parte di quello dei servizi), alle persone più fragili e più in difficoltà, perché la nostra rete di ammortizzatori sociali non è sufficientemente ampia e universale; quindi, interventi ancora emergenziali, sì, ma fortemente selettivi, come primo ingrediente. Un secondo ingrediente è il rilancio veloce di investimenti pubblici e privati per attivare quel moltiplicatore fiscale. Il terzo: riforme che permettano a quei soldi di creare crescita sostenuta, sì, ma anche sostenibile sul piano ambientale e sociale e una crescita inclusiva, perché un Paese ad alto debito come il nostro dovrebbe sapere che senza riforme i soldi da soli non bastano. Per farlo abbiamo bisogno di velocità dei tempi e di coraggio delle scelte. Questo è il momento delle scelte e di priorità chiare. Giustamente, in questi giorni di dibattito parlamentare ci siamo soffermati un po' sul libro dei sogni: è giusto sognare, quando parliamo di linee guida di interventi così importanti, però adesso dovremo passare velocemente all'elenco della spesa la nostra responsabilità politica è fare in modo che esso non sia del tutto sganciato dal libro dei sogni, perché non sappiamo resistere alla porosità delle pressioni categoriali o di *lobby* rispetto alle decisioni vere, alla carne viva della spesa pubblica. Sarebbe un errore politico, se l'elenco della spesa non parlasse al libro dei sogni, e perché queste due realtà si parlino dobbiamo mettere in campo un forte senso di responsabilità verso i giovani e il futuro, neanche il coraggio delle scelte. L'espansione fiscale che votiamo oggi e quella che l'Unione europea ci permetterà avranno un senso solo se non smarriremo la bussola che Governo e Parlamento hanno iniziato a darsi nel dibattito di queste settimane: una crescita sostenibile, ma anche - torno a sottolinearlo - sostenuta, perché questo Paese ha bisogno di rimettersi a correre. Non riusciremo a farlo, com'è stato detto nel dibattito di questi giorni, se non agiremo con forza su tre volani di crescita: l'occupazione femminile, quella giovanile e la ripresa della produttività dei fattori, permettendo al nostro sistema produttivo di agganciare le transizioni tecnologica ed ecologica e rilanciando un percorso di investimenti pubblici. L'occupazione femminile e giovanile non costituiscono soltanto priorità di inclusione sociale, ma sono fattori di crescita.

Si tratta magari di donne che hanno smesso di lavorare perché avevano un contratto temporaneo o perché solo su di loro ricade il peso di provvedere alla cura dei nostri anziani

Senza i sogni, i talenti e le ambizioni di queste donne e di queste giovani, semplicemente, l'Italia non tornerà a crescere. I soldi

Signor Presidente, onorevole Vice Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghe e colleghi,

con una previsione a fine anno del 9 per cento del crollo del prodotto interno lordo e quasi 1.650 miliardi di euro di prodotto interno lordo a seguito di questa riduzione.

del 2,5 per cento nel 2023, con la difficoltà in questo momento di fare delle stime. Ci rendiamo conto Grazie,

efficaci. C'è una prima critica che vorrei rivolgere. Si è discusso tanto di Next generation EU,

relazione ai fondi strutturali che abbiamo a disposizione da anni e senza calcolare la quota di fondi nazionali con cui sono state finanziate delle opere.

Rendiamoci conto che ci sono temi accennati, o comunque sviluppati, che però hanno la natura del manifesto. più che mai di fronte al libro della speranza e lo dico non in senso ironico. Parlo di libro della speranza perché, a oggi, non sappiamo quando passerà la pandemia,

sul nostro prodotto interno lordo, sulle nostre esportazioni e sulle nostre movimentazioni di persone? Che tipo di accordo si concluderà tra la signora Merkel e i Paesi frugali? Permettetemi di aggiungere un'altra considerazione: che effetto avrà

con le normali Note di aggiornamento, in una struttura di economia ferma e stabile e, quindi, con una situazione abbastanza prevedibile.

I fondi dell'Unione europea si dividono in sovvenzioni e finanziamenti: credo che debba essere fatto un grande sforzo da parte del nostro Paese per utilizzare prioritariamente

abbiamo collocato dei BTP triennali a meno di zero e la collocazione BTP triennali a meno di zero significa che non c'è inflazione, che non si cresce, che non c'è pressione della domanda rispetto all'offerta e questo non è un bel segnale quando si parla di ripresa e di espansione. Da parte nostra ribadisco la più completa collaborazione come contributo di idee, ma naturalmente vorremmo una conseguente

Nel corposo documento che è all'esame del Parlamento e che oggi sarà sottoposto al voto, c'è meno di mezza paginetta sulle politiche familiari, tra l'altro da dividersi con le politiche sociali: politiche Ancora una volta si confondono due politiche, due azioni di Governo che in teoria andrebbero, al contrario, nettamente distinte perché un conto sono le politiche sociali, che riguardano la lotta alla povertà, l'inclusione sociale e altre mille cose, un altro sono le politiche familiari, che dovremmo cominciare a considerare come strategiche. Tutto il resto del documento, ricchissimo, corposissimo, con mille voci, non prende in esame il punto di vista fondamentale della prospettiva demografica. Ho sentito tante volte in quest'Aula richiamarsi alla prospettiva demografica, ma in questo documento ce n'è ben poca traccia. Cosa significa cominciare a guardare Significa cominciare a pensare che noi potremmo costruire anche le migliori infrastrutture, potremmo anche fare la migliore *green economy*, potremmo realizzare tutto l'*empowerment* femminile oppure arrivare alla perfezione delle politiche del lavoro, ma se non ci saranno più italiani perché non saranno più venuti al mondo bambini, tutto questo non servirà assolutamente a nulla. Dobbiamo cominciare a entrare nell'ordine di idee che le politiche familiari non sono un accessorio, non sono qualche cosa da da dimenticare o da lasciare per ultimo o su cui spendere due euro alla fine del conto giusto perché, altrimenti, qualcuno fa sentire la sua voce, ma sono le vere politiche strategiche del nostro Paese. Sono le vere politiche su cui concentrare tutta l'attenzione e tutte le risorse del nostro Paese,

un *gap* significativo tra il tasso di figli desiderati dalle famiglie e il tasso di figli concretamente poi avuti. Si tratta di un *gap* significativo. Le Le famiglie vorrebbero almeno due o tre figli mentre, molto spesso, si ritrovano costrette, da ragioni economiche, dalle ragioni di accoglienza sociale della maternità e della paternità, a metterne al mondo uno solo. Quindi, se noi potessimo la possibilità di mettere al mondo i figli che vorrebbero già oggi mettere al mondo, senza alcuna ulteriore promozione se non semplicemente quella di aiutare le famiglie a fare quello che vorrebbero fare,

Certo, siamo ancora lontani dal tasso di rinnovamento, che deve essere comunque superiore al 2; quindi, stiamo comunque parlando di una società in declino, ma almeno sarebbe un segnale concreto. Per fare tutto questo, però, è necessario cambiare la mentalità cambiare la mentalità e io, di questo cambio di mentalità, nelle quattro righe striminzite presenti nella Nota di aggiornamento al DEF non trovo assolutamente nulla. Non c'è alcun cambio di mentalità. Si cerca, invece, ancora di applicare ricette vecchie, che hanno già dimostrato di non funzionare. Non possiamo pensare di dare speranza ai milioni di giovani che vorrebbero sposarsi oppure alle milioni di giovani famiglie che vorrebbero mettere al mondo nuovi figli semplicemente proponendo politiche di sussidio, politiche di sussidio, che nascono dalla stessa sciagurata mentalità che pensa di risolvere i problemi dell'Italia con il reddito di cittadinanza. Non possiamo pensarla in questo modo. Dobbiamo investire su queste famiglie con una forma di fiscalità che finalmente sia premiale. Cerco di spiegarlo ancora più semplicemente: se noi tassiamo nell'ordine del 48 per cento il reddito dei due genitori e poi, graziosamente, restituiamo quattro soldi sotto forma di assegno oppure di sussidio, non stiamo dando affatto speranza alle famiglie. Anzi, stiamo sostanzialmente deprimendo la speranza di vita la speranza familiare, ma stiamo anche deprimendo l'economia di questo Paese. Qual è invece la politica che la Lega sta proponendo da tempo e che, su questo punto, ha già dato prova di funzionare in alcuni ristretti ambiti in cui si è riusciti ad applicarla? La politica deve essere quella della *no tax area*. I carichi familiari non debbono cioè essere tassati, perché, se c'è un padre che ha un reddito di 50.000 euro l'anno ma ha tre figli, quel padre non deve veder tassato neppure un euro dal suo reddito, perché con 50.000 con 50.000 euro l'anno e tre figli, si fa fatica ad arrivare alla fine del mese. *(Applausi)*. E mi metto nei panni degli operai che, con molto meno di 50.000 euro all'anno e magari tre, quattro o cinque figli, riescono comunque a sbarcare il lunario. Veramente a loro va tutta la nostra stima, perché oggi mettere al mondo un figlio in Italia è un atto da eroi, è un atto eroico. Dicevo che bisogna uscire dalla mentalità del sussidio ed entrare finalmente nella mentalità della politica familiare di natura fiscale. Questo avrei voluto leggere nella Nota di aggiornamento al DEF e invece cosa trovo? Trovo il *family act*, trovo il piano strutturale integrato di politiche familiari, che in realtà non ha neppure un euro Quindi di cosa stiamo parlando? Di un sogno, di una pia illusione che tuttavia non vede spostato neanche un euro nelle previsioni di spesa. Questa volta non potrete nascondervi dietro alla solita fandonia del fatto che non ci sono soldi, perché - guarda un po' - i soldi questa volta ci sono, ci sono eccome. Vogliamo allora mettere alla prova le buone intenzioni di questo Governo e vogliamo vedere se davvero si vogliono fare politiche familiari o se ancora una volta si vuole raccontare qualche menzogna e qualche leggenda metropolitana. Fare politiche familiari, come vi dicevo, significa cambiare mentalità. La *no tax area* è costruita in modo molto semplice: ogni figlio e ogni persona a carico (che può essere anche un anziano, un disabile o una persona che ha bisogno di cura)

Deve essere calcolato il reddito dell'intero nucleo familiare e poi, sulla base di quello, devono essere fatti i conti e là si deve andare a estrapolare, per ogni figlio a carico e per ogni carico familiare, una *no tax area*, che può essere ovviamente variabile in base alla situazione ma su quella entrata non debbono essere pagate tasse. Voi lo sapete che oggi in Italia i bambini pagano le tasse prima ancora di nascere? Ciascuno di voi credo abbia avuto il piacere di fare un piccolo regalo a qualche bambino che ancora non era nato, perché magari figlio di amici in attesa; quando c'è una donna incinta, si va a trovarla e magari si porta un vestitino o qualcos'altro. Tutti voi avete pagato l'IVA tutti voi avete pagato un imposta sul valore aggiunto su quel prodotto; cioè noi paghiamo tasse, siano esse dirette o indirette, prima ancora di venire al mondo. La prima cosa che mi hanno dato quando sono nati i miei tre figli non è stato un semplice regalo, una pacca sulla spalla, un sorriso, un dire: «Bravo, hai messo al mondo tre figli, che poi pagheranno le tasse e pagheranno le pensioni a tutti gli italiani»;

modificata e potrebbe diventare qualcosa di più favorevole verso la vita nascente. Ho concluso, signor Presidente.

Lo ripeto: il miglior investimento che oggi l'Italia possa fare è quello di mettere latte, possibilmente esentasse, nei biberon.

onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, ricordo quando lo scorso anno discutevamo questo stesso documento programmatico in quest'Aula, tra questi banchi; mai avremmo pensato che sarebbe stata scritta una pagina di storia così difficile. Dopo quello cui abbiamo assistito negli ultimi dieci mesi, ciò di cui parliamo oggi ci appare una lingua veramente difficile da tradurre. Non solo il nostro Paese, ma l'Europa e il mondo intero hanno vissuto uno sconvolgimento senza precedenti. Sebbene la presente Nota di aggiornamento si riferisca al triennio 2021-2023, il Governo ha anche elaborato proiezioni macroeconomiche e di finanza pubblica a sei anni, che costituiranno la base sia per valutare gli impatti del programma di investimenti e degli altri interventi finanziati dal Next generation EU sia per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di notare negli ultimi mesi, non è assolutamente facile interpretare il futuro. Proprio per questo motivo è ancor più grande la responsabilità che, come Governo e come maggioranza, ci stiamo assumendo per traghettare il nostro Paese fuori da questo pantano pandemico. Lo traghetteremo con la fiducia che ne usciremo uniti, aiutandoci reciprocamente, forse ansimanti, sì, ma salvi. Quello che chiediamo però - specifichiamolo - non è una fiducia incondizionata verso le decisioni prese, ma un sentimento di unità nazionale che deve prevalere sui particolarismi e sulle decisioni unilaterali. Del resto, la storia è ricca di momenti difficili dai quali l'umanità è sempre uscita più forte di prima. Ciò che è diverso rispetto al passato è la ferrea volontà di uscirne tutti insieme. Nelle pandemie una volta sopravvivevano solo i più forti o i più fortunati; oggi è nostro compito e dovere salvaguardare ogni singola vita umana. Il Governo può - e lo sta facendo - alleviare gli effetti di ogni perdita economica o difficoltà lavorativa. Purtroppo, ciò che non possiamo fare è restituire la vita ai tanti che ci hanno lasciato e che meritano di essere l'anima stessa del nostro operato, responsabile e prudente, dei prossimi mesi. prossimi mesi. La NADEF contiene al suo interno lo spirito di un'Europa unita e solidale. Lo scenario macroeconomico in essa tracciato contiene tutti gli strumenti che saranno messi a disposizione del nostro Paese con il piano Next generation EU e in particolare che saranno destinati ai progetti inseriti nel Piano nazionale per la ripresa la residenza all'inizio del prossimo anno. Le risorse che dovrebbero essere attribuite all'Italia sono stimate in circa 205 miliardi, di cui 78 di sovvenzioni e fino a 127 di prestiti. La prossima legge di bilancio e le sovvenzioni del *recovery and resilience facility* avranno un valore complessivo pari a circa il 2 per cento del PIL nel 2021; l'obiettivo prioritario sarà valorizzare questi capitali, al fine di garantire la riduzione dell'impatto sociale ed economico della crisi pandemica, sostenendo innanzitutto il reddito dei lavoratori, nonché l'occupazione. In tal senso occorre sottolineare come le misure fino ad ora adottate abbiano consentito di scongiurare gli scenari più avversi. L'introduzione di strumenti quali la cassa integrazione in deroga ha fatto sì che la percentuale di occupati sia scesa in misura di gran lunga inferiore alla caduta dell'*input* di lavoro legato alla chiusura delle attività produttive. L'Istat rileva un incremento congiunturale dell'occupazione dello 0,4 per cento, sia nel mese di luglio che nel mese di agosto scorsi; peraltro, le recenti manovre di stimolo dell'economia intraprese con il cosiddetto decreto rilancio e con i successivi provvedimenti hanno comportato una variazione in positivo al 5,1 per cento della previsione di crescita economica per il 2021 rispetto alle precedenti stime del DEF che si attestavano al 4,7 Stiamo lavorando attivamente nelle Commissioni parlamentari proprio per strutturare un piano di interventi per un efficace utilizzo dei fondi europei. Verranno rilanciati gli investimenti pubblici e privati e attuate importanti riforme all'interno di un disegno di rilancio e di transizione verso un'economia più innovativa, più sostenibile dal punto di grazie a tutto un grande piano di riforme basato sull'impulso statale in tutti i settori strategici del nuovo millennio. Nessun settore economico verrà lasciato indietro (certamente non si vuole investire per tornare indietro); l'obiettivo è accompagnare la ripresa guardando a scenari futuri. Questo piano non è una scatola chiusa ed ermetica, ma aperta a suggerimenti e a contributi da parte di tutte le rappresentanze. Vogliamo che si inneschi un dialogo positivo, non strumentale a critiche sterili e viziato da preconcetti Dagli imprenditori arrivano quotidianamente stimoli a supportare la ripresa con interventi sul costo del lavoro ed è proprio nell'interesse del Paese una riforma strutturale che riduca la tassazione sul lavoro e che incida positivamente sui redditi medi, da sempre la fascia più ampia della popolazione lavorativa, senza però dimenticare anche tutti coloro che invece hanno redditi più bassi e sono stati duramente colpiti dalla crisi. Sappiamo bene che il settore industriale può essere la vera locomotiva della ripresa occupazionale, è certo che, seppure il Governo fornirà il propellente per avviare questo motore, poi saranno gli imprenditori stessi ad avere l'onere di non tenere il freno a mano tirato, come troppo spesso è successo in passato. Si prospetta anche una manovra di bilancio imponente, intorno ai 40 miliardi, con un rapporto di finanziamento in *deficit* di oltre 22 miliardi di euro, cui si affiancherà però una scrupolosa gestione della finanza pubblica volta a ridurre l'indebitamento netto della pubblica amministrazione, compatibilmente con la riduzione del rapporto debito-PIL.

Si delinea così un piano progressivo di rientro, tale da ricondurre il debito della pubblica amministrazione al di sotto del livello pre-Covid-19 entro la fine del decennio. Gli indicatori congiunturali ci danno ragione, segnalando nel complesso un andamento positivo e di graduale ripresa dell'economia, che speriamo si traduca in una maggiore fiducia delle famiglie e del settore produttivo, nonché nell'aumento della domanda globale. La fiducia si guadagna lentamente, passo dopo passo, mattone dopo mattone; non l'abbiamo mai data per scontata, e sappiamo molto bene che basta una piccola crepa per rovinare tutto in un istante. Ma il lavoro, se buono, è giusto che venga messo in risalto senza preconcetti, con l'auspicio di una rigogliosa rinascita dopo questo rigido inverno.

ora che siamo di fronte a un crocevia importante con la NADEF e con gli altri provvedimenti che ci aspettano, mi preme ricordare a questa Assemblea alcuni aspetti che riguardano la base del successo del *recovery fund.* Qui, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo ribadito in maniera netta e decisa che a fare la differenza saranno i settori di intervento. Il grido di dolore del nostro tessuto produttivo continua a farsi sentire in questo difficilissimo 2020, segnato in maniera durissima dal coronavirus e che ci è costato tantissimo in termini di PIL e di economia reale. Per questo, tutti i nostri comparti produttivi ci chiedono uno sforzo mai visto per dare loro non solo risposte decise inerenti all'emergenza, ma anche tutti quegli accorgimenti strutturali che le nostre piccole e medie imprese attendono da anni. A tal fine, già le linee guida sul *recovery plan* che abbiamo tracciato parlano chiarissimo. Le stelle polari da seguire sono quelle della digitalizzazione e dell'innovazione, dell'istruzione e della formazione, della rivoluzione *green* e della transizione ecologica, della mobilità buona e dell'equità sociale, della tutela della salute e di una sanità pubblica che abbia le risorse che merita, e non i rimasugli delle diverse leggi di bilancio, come accaduto per almeno due decenni. Sforzi da parte della politica, quindi, ma anche buona volontà ad esempio da parte dei nostri amici di Confindustria. Io stesso in prima persona ho fatto mie delle proposte legislative che trovo necessarie per supportare comparti industriali strategici per il nostro Paese. Ma quello che non vedo nella presidenza attuale è la volontà di collaborare costruttivamente. Il Governo e il Parlamento hanno certamente il dovere di supportare la ripresa con strumenti legislativi, ma è altrettanto necessario superare la storica resistenza degli imprenditori italiani agli investimenti in risorse umane e in ricerca e sviluppo; investimenti che non seguiranno tra tre o quattro anni, poiché servono subito. Per le nostre imprese lo sforzo che serve è suppletivo. Da questa pandemia il nostro tessuto produttivo dovrà uscire rinfrancato e consapevole che lo Stato non è un nemico dell'iniziativa privata, ma un prezioso alleato pronto a concorrere perché il nostro Paese, seconda manifattura d'Europa, torni ai livelli produttivi che merita. merita. È mossa da questo obiettivo una misura epocale come il superbonus al 110 per cento: un meccanismo fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle per produrre un vero e proprio *shock* in un comparto cruciale per la nostra economia e ad altissimo moltiplicatore economico come quello dell'edilizia. Un'edilizia che vogliamo diversa: più sostenibile, virtuosa e all'avanguardia. Inserito nel decreto-legge rilancio, già nel cosiddetto decreto-legge agosto il superbonus è stato perfezionato e ne è stata ampliata nei fatti la platea; ora va ulteriormente consolidato, perché si tratta di un ampio piano di interventi di ristrutturazioni energetiche ed antisismiche che, a detta di tutte le principali associazioni imprenditoriali, da Confindustria all'ABI, da Unioncamere all'ANCE, passando per le associazioni professionali, è in grado di imprimere una netta inversione di tendenza a un settore che ha tribolato molto, ma che va sostenuto e aiutato. Questa novità può creare centinaia di migliaia di posti di lavoro. Non è un nostro pronostico, ma il risultato di proiezioni concrete. Non solo il superbonus è da irrobustire, come maggioranza abbiamo convenuto sulla necessità di arrivare alla stabilizzazione - almeno su base triennale - di transizione 4.0, da noi già trasformata e semplificata nella scorsa legge di bilancio. Potenziare queste misure è quanto di più ragionevole si possa fare per dare davvero un contributo concreto alla nostra industria. In questo caso, facciamo riferimento a quel massiccio pacchetto di incentivi fiscali, già oggi del valore di 7 miliardi di euro l'anno, che permetteranno alle imprese di investire in beni strumentali, macchinari, beni tecnologici, *software* e tutto ciò che consentirà loro di competere al meglio sui mercati interni e internazionali. C'è poi un capitolo a parte che va affrontato, in cui si fa riferimento al tessuto produttivo del nostro Paese, che riguarda la valorizzazione della capacità produttiva del Meridione.

Spalmata su base pluriennale, tale misura permetterà investimenti più massicci e duraturi nelle Regioni meridionali, con un impatto occupazionale di tutt'altra molla rispetto a quella attuale. Il Sud può davvero diventare il simbolo della rinascita del nostro Paese nel *post-*Covid. Dobbiamo farci trovare pronti quando sarà il momento. Il percorso che stiamo facendo per arrivare alla legge di bilancio deve muoversi seguendo questa strada. C'è tanto altro ancora da affinare per le nostre piccole e medie imprese. Con il Governo stiamo lavorando a spron battuto nel segno della concretezza: dal commercio all'industria, dall'agricoltura al turismo, dalla logistica all'artigianato. Le risposte da dare sono moltissime, ma il coraggio, le proposte e le idee ci sono. La strada è tracciata. Il Covid, purtroppo, è destinato a colpire ancora le nostre imprese. Queste ultime sanno che il Governo e la maggioranza in Parlamento saranno sempre al loro fianco, pronti allo sforzo massimo per non far morire la produttività nel nostro Paese.

intervengo solo per una precisazione. Abbiamo visto che l'elenco degli iscritti, rispetto a quanto era previsto alla ripresa dei lavori, si è improvvisamente allungato. La domanda è: di solito ci viene detto viene detto che la possibilità di iscrivere le persone a parlare deve essere data prima dell'inizio della seduta. Capisco che possa esserci anche tempo a disposizione, però è possibile che questo si

non ha i 161 voti necessari per approvare lo scostamento di bilancio, lo faccia sapere alle opposizioni, lo dica chiaramente e lo dica soprattutto al Paese.

Il Presidente del Senato ha accolto tale richiesta e quindi sono stati inseriti, nell'ordine in cui è stata presentata

Signor Presidente, la discussione odierna sulla NADEF si lega inevitabilmente al percorso già intrapreso per far fronte all'emergenza un percorso che parte dal decreto cura Italia e prosegue con i decreti liquidità, rilancio, semplificazioni e agosto e passa adesso per la NADEF e l'imminente legge di bilancio, che a sua volta andrà letta in combinato disposto con il *recovery fund.* Non c'è dubbio, come scritto nella NADEF, che un percorso di rilancio del Paese non potrà fare a meno di una profonda e organica riforma fiscale, così come la riforma e la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la velocizzazione dei tempi della giustizia, anche la riforma fiscale sarà decisiva nell'orizzonte di opportunità che ci si apre davanti con il *recovery fund* e con la possibilità - questo occorre valutarlo - di emettere titoli di debito pubblico a tasso zero o negativo, come nel caso, ad esempio, dei titoli a tre anni (è notizia di ieri). Ho sentito dire in Assemblea anche ieri, in modo abbastanza strumentale, che la riforma fiscale non c'è e che non se ne vedrà traccia prima di qualche anno. La riforma fiscale sicuramente non può essere scritta in emergenza e non può essere scritta in poche settimane. Occorre avviare la discussione, come sta facendo il Governo. Occorre rendere su questo do ragione all'opposizione. Questo lo si può fare anche con una legge delega, di cui lo stesso Governo peraltro ha parlato. La riforma fiscale è un percorso, per affrontare il quale bisogna comunque partire. L'anno scorso abbiamo tagliato il cuneo fiscale per 16 milioni di contribuenti, ai quali adesso in manovra confermeremo quel taglio, che valeva fino alla fine del 2020. Stiamo lavorando per inserire nella manovra l'assegno unico familiare, legato all'ISEE, che ci permetterà di razionalizzare tutta una serie di bonus e agevolazioni, oggi eccessivamente polverizzata. Dalla NADEF emerge il numero effettivamente

La pressione fiscale, nei prossimi anni, è data in riduzione a legislazione vigente e a maggior ragione scenderà con le misure che andremo a implementare. L'uso della tecnologia sarà fondamentale, sia per semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadini, sia per contrastare, in funzione preventiva, un'evasione fiscale, che in Italia raggiunge livelli ancora troppo alti. alti. Credo che dovremmo parlare proprio di funzione preventiva ovvero di prevenzione dell'evasione, perché abbiamo visto che il termine «lotta» all'evasione purtroppo non ha funzionato negli ultimi anni e ha contribuito a creare un clima di sfiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente. Il Governo questo lo sa e lo abbiamo potuto vedere tutti con l'introduzione della fatturazione elettronica. L'evasione si previene con la tecnologia. La fine del percorso sarà la ricalibratura dell'Irpef, che dovrà sensibilmente alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, quello più penalizzato, soprattutto a causa del salto di 11 punti dall'aliquota del 27 per cento a quella del 38 per cento. Parliamo quindi di un percorso, non di ritardi o di libri dei sogni, come abbiamo sentito. abbiamo sentito. Si parla di collaborazione tra maggioranza e opposizione: l'opposizione chiede di essere coinvolta - e sono d'accordo - a patto che ci sia la consapevolezza che dobbiamo essere veramente uniti nell'affrontare lo sforzo. Poi però sento una parte dell'opposizione, ancora ieri in Aula, diffondere strumentalmente falsità, come il fatto che il Governo starebbe cancellando quota 100, quando la stessa Lega al Governo ha convenuto di varare la misura come triennale e quindi con scadenza a fine 2021. poi dire che il Governo starebbe cancellando opzione donna, quando già ieri, quando il senatore Salvini l'ha detto, tutti sapevamo che il Governo aveva deciso di prorogarla nella manovra di bilancio. O ancora, sentiamo dire che l'INPS non sta pagando le casse integrazioni, quando tutti sappiamo che ai primi di settembre l'INPS ha pagato 11,06 milioni di casse integrazioni su 11,4 milioni: la percentuale mi sembra abbastanza elevata e difendibile. Dico ciò perché mi chiedo se vi sia l'effettiva volontà di collaborare da parte dell'opposizione. Mi auguro comunque che tutti possano davvero partecipare a questo sforzo, anche condividendo soluzioni innovative. Come MoVimento 5 Stelle ne abbiamo diverse: il superbonus, non mi stancherò mai di dirlo, è una nostra misura e dobbiamo dirlo noi per primi. ideata e voluta dal MoVimento 5 Stelle. È stato introdotto il principio della libera circolazione dei crediti d'imposta, allargato anche ad altre forme di agevolazione fiscale. Si tratta adesso di fare un ulteriore passo in avanti e di consentire l'utilizzo di questi crediti come mezzi di pagamento di beni e servizi, una volta certificati su una piattaforma informatica, in sicurezza e nel rispetto di tutti i vincoli. Presidente, oggi siamo qui a confrontarci sulla possibilità di progettare il Paese del futuro. È merito di questo Governo e della maggioranza, in cui un ruolo decisivo è e continuerà ad essere svolto dal MoVimento 5 Stelle. Al Governo chiedo maggiore coinvolgimento del Parlamento, della maggioranza e dell'opposizione. All'opposizione, ad una certa opposizione, chiedo di non farsi portatrice di solo rancore.

definisce il perimetro di finanza pubblica entro cui si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2021-2023. Gli interventi dovranno essere rivolti a sostenere nel breve termine, per tutta la durata della crisi Covid-19, i lavoratori nei settori produttivi più colpiti, a valorizzare appieno le risorse messe a disposizione dal programma Next generation EU, per realizzare investimenti e riforme di portata e profondità inedite, a rafforzare gli investimenti a sostegno della ripresa nel Mezzogiorno e delle aree interne per migliorare la coesione territoriale. Saranno poi rivolti ad attuare un'ampia riforma fiscale che migliori l'equità, l'efficienza e la trasparenza del sistema tributario, ad assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini, dell'equità e della produttività dell'economia; infine, saranno volti a ricondurre l'indebitamento netto della pubblica amministrazione verso livelli compatibili con una costante e significativa riduzione del rapporto fra debito e PIL. Un programma ambizioso, in cui non può mancare l'obiettivo della coesione territoriale. L'annosa questione dello spopolamento delle aree interne, siano esse montane o insulari, è un problema mondiale. Abbiamo inaugurato il terzo millennio con un primato che deve far riflettere: la popolazione mondiale che vive nelle metropoli e nelle megalopoli ha superato quella che vive nel resto del pianeta; continuando di questo passo, arriveremo ai due terzi, poi ai tre quarti e così via. Ma è accettabile una situazione simile? È compatibile con l'ecosistema, con una dignitosa esistenza umana? Da tempo vari decreti-legge e iniziative legislative annunciano interventi volti a contrastare tale situazione, senza che venga fatta la scelta politica di riservare risorse capaci di invertire questa tendenza. Ora i soldi ci sono e non possiamo permetterci di perdere l'occasione per la riqualificazione dei borghi e dei paesi, per opere infrastrutturali, per il mantenimento e il rafforzamento dei servizi pubblici essenziali (scuole, presidi sanitari, posti di pubblica sicurezza, prima di ogni altra cosa), per trasporti più adeguati e connettività attraverso la banda larga. È così che si contrasta lo spopolamento. Con riferimento allo scenario macroeconomico internazionale, constatiamo con preoccupazione come nella prima metà del 2020 l'economia mondiale abbia registrato la battuta d'arresto più profonda dalla Seconda guerra mondiale e ciò in conseguenza del diffondersi della pandemia da Covid-19. Nonostante le misure straordinarie di politica fiscale e monetaria per sostenere i redditi dei lavoratori e il tessuto produttivo, adottate dai Governi e dalle banche centrali, il blocco produttivo ha determinato una contrazione del PIL e del commercio mondiale a livelli *record* e lo scenario globale appare orientato ancora al ribasso, in ragione del fatto che all'evoluzione dell'epidemia nel mondo - che in molti Paesi continua a manifestarsi con particolare intensità - si affiancano rischi connessi a tensioni geopolitiche preesistenti all'epidemia e acuitesi di recente: dai rapporti commerciali tesi tra Stati Uniti e Cina, alle difficoltà del processo di negoziazione della Brexit, fino all'emergere di nuove complicazioni nei rapporti fra Turchia e Russia. Come molti interventi in quest'Aula tra ieri e oggi hanno messo in evidenza, la geopolitica del Mediterraneo è completamente mutata. Al posto della cooperazione bilaterale, multilaterale e decentralizzata, assistiamo all'*escalation* delle guerre per procura, che rendono particolarmente fragili gli equilibri faticosamente costruiti nel ventennio precedente. La politica estera del nostro Paese non può ridursi alle pur giuste misure a favore del *made in Italy* attraverso il rifinanziamento del fondo rotativo per l'internazionalizzazione di enti fieristici e delle *start-up* innovative. Occorre rilanciare la dimensione mediterranea dell'Unione europea e il suo ruolo attivo per la pace e la promozione dei diritti umani. *(Applausi)*.

Governo, onorevoli colleghi, in questa Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza per il settore sanitario si riprende la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea a rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario, migliorando la *governance* e la capacità di risposta alle crisi, per colmare quella carenza di investimenti pubblici che ha colpito il settore sanitario. Abbiamo ripetuto più volte in quest'Assemblea come negli ultimi dieci anni siano stati tagliati 37 miliardi di euro dal settore pubblico; abbiamo perso 71.000 posti letto, soprattutto nelle aree critiche, tra cui quelli di terapia intensiva; 46.000 operatori (medici e infermieri) hanno lasciato il servizio sanitario pubblico per veder riconosciuto il proprio merito in strutture private.

Già nella scorsa legge di bilancio abbiamo stanziato 2 miliardi di euro per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico dei nostri ospedali. Avevamo depositato un emendamento a nostra firma, che prevedeva di destinare il contributo previsto per i medici di medicina generale per dotarsi di strumenti diagnostici proprio all'acquisto di strumenti di telemedicina. Quanto sarebbero stati utili questi strumenti di telemedicina a disposizione dei medici di medicina generale anche nella gestione di questa pandemia! Abbiamo puntato sulla digitalizzazione perché, per noi, la cartella clinica elettronica e il fascicolo sanitario elettronico devono diventare realtà in tutte le Regioni italiane. Nelle nostre riforme puntiamo sulla ricerca e l'Italia è il Paese in cui si investe di meno in ricerca e sviluppo ed è il Paese che ha il numero più basso in Europa di ricercatori per numero di abitanti.

ente di ricerca pubblico italiano, so bene quanto sia mortificante non avere a disposizione dei fondi destinati a progetti di ricerca. Abbiamo puntato sulla valorizzazione degli operatori sanitari, a partire dalla loro formazione. Si parla di imbuto formativo, che si è creato perché non si è saputo programmare: non c'è stata una programmazione degli degli specialisti nel settore sanitario in base al fabbisogno di salute della popolazione. Per questo nella scorsa legge di bilancio abbiamo stanziato 3 milioni per

che servirà proprio a programmare il fabbisogno di specialisti. Non c'è una carenza di medici, ma di specialisti in alcuni settori. Bisogna valorizzare il personale anche stabilizzando i precari della sanità. Sappiamo tutti che se il Servizio sanitario nazionale ha retto all'onda d'urto è per la resilienza e la dedizione di tutti gli operatori sanitari, molti dei quali, a causa del blocco delle assunzioni in sanità, che finalmente abbiamo superato, lavorano da decenni con contratti precari. (*Applausi*). Abbiamo pertanto stabilizzato un primo blocco di precari e proseguiremo in questo percorso. Abbiamo puntato su una riforma della *governance*, a partire dalle nomine dei dirigenti e dei direttori generali, che per noi devono essere meritocratiche e non per appartenenza politica, mettendo sempre al centro il merito e le competenze. Rivedere la *governance* significa anche rafforzare il ruolo di indirizzo dello Stato centrale perché non possiamo più permetterci un diverso accesso alle cure dei cittadini sul territorio nazionale. Rivedere la *governance* implica una revisione del rapporto tra sanità pubblica e privata, con la sanità pubblica che deve essere una stampella e non una spugna che assorbe risorse fondamentali per il servizio pubblico. Rivedere la *governance* significa anche rivedere l'accesso ai farmaci e alle cure. I farmaci devono essere sempre più innovativi e personalizzati. Nella scorsa legge di bilancio abbiamo stanziato un miliardo di euro per i farmaci innovativi. Abbiamo previsto dei nuovi metodi di rimborso del costo del farmaco

Rivedere la *governance* significa attuare finalmente quel Piano nazionale cronicità, che in realtà è applicato solo in pochissime Regioni, e riformare totalmente la medicina territoriale, che non è solo medicina generale, ma è rete di cure primarie e cure intermedie. Questi pilastri su cui abbiamo finora lavorato con le nostre proposte di legge ed emendative sono anche i pilastri di questa Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e saranno i pilastri della prossima legge di bilancio. Mettiamo al centro la programmazione in base al fabbisogno di salute della popolazione. Mettiamo al centro le competenze e anche la valutazione dei risultati, cosa che in questo Paese, purtroppo, spesso è un'utopia. Dobbiamo riformare la sanità per renderla veramente strumento di tutela della salute e solo con progetti definiti e solidi useremo al meglio i fondi del *recovery fund* e, in generale, lo strumento del Next generation EU. Abbiamo capito a nostre spese che non serve spendere meno, ma serve spendere meglio riducendo soprattutto sprechi e inefficienze. Non avremo un'altra occasione se non sapremo usare questa tragedia per avere il coraggio di mettere finalmente in atto le riforme che il Paese attende da almeno un decennio.

Signor Presidente, ogni generazione si crede destinata a cambiare il mondo. La mia - scrisse Albert Camus sa che non lo cambierà, ma il suo compito è persino più grande e consiste nell'impedire che il mondo vada in pezzi, in pezzi, erede di una storia avvelenata in cui si mescolano le rivoluzioni fallite, la tecnica impazzita, gli dei morti e le ideologie esauste. Dove poteri mediocri possono oggi annientare tutto, ma non sono in grado di convincere, dove l'intelligenza si è abbassata fino a farsi schiava dell'odio e dell'oppressione, questa generazione ha dovuto in se stessa e intorno a sé ricostruire, partendo dalle sue stesse negazioni, un po' di quello che fa la dignità di vivere e di morire. e di morire. Faccio questa citazione per sottolineare il fatto che non è un caso, come accade in Assemblea in questi mesi, se le discussioni che ci troviamo ad affrontare sui singoli provvedimenti non sono mai limitate solamente ad essi, ma cercano di andare oltre analizzando la realtà che ci corre con i suoi problemi intorno agli occhi e immaginando magari un domani migliore. Sono discussioni sulla grande opportunità di progettare il futuro di questo Paese. Questa enorme occasione passa, come è stato ripetutamente detto in questa Aula, per le ingenti risorse del piano Next generation EU,

dei contributi di tutte le forze politiche. Siamo infatti di fronte ad una crisi epocale e quindi ad una svolta che assorbe tutti gli aspetti dell'esistenza. Questo invito sincero alla collaborazione non è un pretesto da esibire in un discorso in questa sede o in interviste televisive, ma trova l'impegno quotidiano del MoVimento 5 Stelle anche attraverso quello che, per esempio, è successo questa mattina in Commissione finanze dove, dovendo esprimere un parere sulla NADEF, noi come maggioranza abbiamo rivolto alle forze dell'opposizione un invito sincero a analizzare il provvedimento,

della realtà drammatica del Paese, delle esigenze che i cittadini ogni giorno ci manifestano e che il presidente della Repubblica Mattarella non si stanca mai di ricordarci. Mai come in questo momento c'è bisogno della massima unità; in una dialettica anche forte tra le forze politiche, c'è bisogno però di uno spirito di collaborazione costituente e repubblicano, il solo che ci può consentire oggi di risolvere i problemi dei cittadini e creare le condizioni economiche e sociali affinché nei prossimi anni il Paese possa tornare a vivere e correre, socialmente ed economicamente coscienti e cosciente, come io sono, che questa non è una opportunità riservata solo a chi oggi governa. Questa è invece un'opportunità che la maggioranza offre al Paese e all'opposizione, sapendo che, in una nobile e sana e sana pratica dell'alternanza, oggi tocca a noi e domani toccherà a loro, con l'augurio, sin da oggi, che possano fare il meglio per l'Italia.

però avere tutti la consapevolezza che non c'è un domani per cambiare la dialettica parlamentare e lo spirito di collaborazione, che devono essere, appunto, repubblicani. L'occasione passa oggi,

una feroce e puntuale critica all'azione di Governo, ma anche qualche primo timido segnale alla maggioranza affinché si instauri uno spirito di collaborazione. Noi siamo qui

non ci sono le risposte a tutti i problemi e - a mio giudizio - è sbagliato criticare questo o quel punto, questa o quella cifra di previsione su quella che sarà l'economia nel 2021 o nei prossimi anni. Dobbiamo essere coscienti e dire ai cittadini che, alle prese con la pandemia, della quale non vediamo una fine certa, anche le previsioni economiche sono precarie. Quella che è certa è l'azione sincera di questo Governo che, nella

che ogni patto repubblicano e qualsiasi patto sociale si fondano sulla capacità contributiva di dare onestamente. Non si può chiedere a un Governo e a uno Stato di avere sovvenzioni se, poi,

Abbiamo il problema di controllare l'uso delle risorse, a cominciare da quello che fanno i singoli cittadini, ma anche le imprese. Forse, da questo punto di vista, se vogliamo essere un Paese diverso, dobbiamo capire che, se vogliamo iniziare

di attingere all'esperienza tedesca per cercare di coinvolgere, nella gestione... *(Il microfono

Signor Presidente, la Nota di aggiornamento ormai è un esercizio di solfeggio cantato: voi gorgheggiate delle note su un pentagramma scritto dall'Europa, ma all'Europa delle famiglie italiane, non interessa nulla; del resto non è attrezzata per scrivere questa musica qui. Ieri come oggi, il Ministero dell'economia e delle finanze nella sua struttura è un pezzo del sistema di potere, della cabina di regia di un'Europa a sola trazione finanziaria e speculativa. Non c'è, nel suo *radar*, l'interesse delle aziende italiane, delle famiglie italiane, dei lavoratori italiani. La nomina alla presidenza Unicredit di Pier Carlo Padoan, ex Ministro dell'economia e delle finanze di Renzi e Gentiloni, lo conferma. E alla fine arrivò Pier Carlo - potremmo dire - perché prima di lui al MEF ci fu il compianto Fabrizio Saccomanni, Ministro con Enrico Letta; in via XX Settembre arrivò dalla plancia di comando di Bankitalia. Cosa fece Saccomanni dopo l'incarico ministeriale? Andò a ricoprire l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit - ma tu guarda - fino al giorno della morte. Prima ancora di Saccomanni, al Ministero dell'economia e delle finanze c'era Vittorio Grilli: arrivava dei vertici del Tesoro, dove fu a capo della Direzione per le privatizzazioni; poi, tra l'altro, questo incarico lo sospese, perché andò a Credit Suisse - guarda caso vanno sempre nelle banche importanti - salvo poi ritornare un'altra volta al Ministero, dove divenne Ragioniere generale dello Stato, poi Direttore generale del Tesoro e infine Ministro nel Governo Monti. Evviva! Bene, che cosa va a fare Grilli terminato l'incarico al MEF? Va alla banca d'affari J.P. Morgan come presidente *corporate* area Europe, Medio Oriente e Africa. Evviva! Finita? No, ne abbiamo ancora uno da servire. Si chiama Domenico Siniscalco, per gli amici Mimmo. Mimmo arrivò a ricoprire l'incarico di Ministro dell'economia dalla Direzione generale del Tesoro, dove aveva preso il posto di Mario Draghi, il quale - si sa - fece i bagagli per andare in Goldman Sachs e poi ritornare in Banca d'Italia e alla BCE. Ora vedremo se lo faranno Presidente della Repubblica e Dio non voglia. Bene, cosa andrà a fare anche Mimmo Siniscalco una volta lasciato il Ministero? Va a fare il vice presidente *international* di Morgan Stanley e a ricoprire altri incarichi non meno importanti. Tutto questo *exscursus* ci fa capire che il MEF è una delle più strategiche e funzionali sale macchine del sistema: arrivi se se ne fai parte e se ne accetti le regole. Il MEF serve per il sistema, non per l'economia reale, per le famiglie e per i lavoratori. Da quando siamo entrati nelle logiche europee, lo è ancora di più e anche questa Nota di aggiornamento a questi incastri di giochi finanziari, dove al popolo lasciate le briciole, vendendole come un successo e i dati lo dimostrano: nove milioni di cartelle esattoriali e medie imprese e famiglie, imprese non pagate dalla pubblica amministrazione; regole sempre più assurde nel settore della ristorazione, dell'artigianato, del commercio; sistema del credito lontano anni luce dalle imprese; pressione fiscale inversamente proporzionale, politiche elusive per le multinazionali

famiglie sono impaurite, stressate dalla crisi e dalle sue evidenti ingiustizie sociali; le bollette della luce e del gas sono vergognose, perché non avete il coraggio di togliere gli oneri di sistema. Altro che *new green deal*! Le bollette vanno drasticamente ridotte, e non di qualcosina con le forbicine, perché le famiglie italiane ne hanno le tasche piene. Ma a voi che interessa? Tanto le preoccupazioni del Governo sono di dare a Unicredit presieduta da Padoan quella Montepaschi che l'ex ministro Padoan aveva nazionalizzato. Il solito Governo amico degli amici! Quindi: viva l'Italia, onore agli italiani e via dall'Europa. Viva Italexit!

Sono, inoltre, pervenute alla Presidenza, sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, le proposte di risoluzione nn. 1, presentata dai senatori Marcucci, Perilli, De Petris, Faraone e Unterberger,

nella mia replica cercherò di indirizzarmi verso alcuni punti sollevati dai miei colleghi nei loro interventi. Ritengo, infatti, opportuno che, in questa sede, si faccia chiarezza. Si deve far sì che chi ci segue possa avere informazioni corrette e depurate dalle posizioni politiche. I dati, insomma, devono essere dati e non devono essere distorti per un vantaggio politico. *In primis*, in merito alla questione del recupero degli importi da parte del Governo, ritengo che non sia corretto quanto affermato dalla senatrice Toffanin, e cioè che si userà il recupero dell'evasione fiscale. È certamente vero che il Governo continuerà a perseguire politiche di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale e, in generale, di miglioramento della *compliance*, che negli ultimi anni hanno conseguito risultati notevoli, superiori alle aspettative, ma le proiezioni programmatiche non includono ulteriori aumenti del gettito derivanti dal contrasto all'evasione. Si prevede, invece, la costituzione di un fondo, da alimentare con le entrate effettivamente generate da tale attività, che sarà destinato al finanziamento di interventi di riforma fiscale e alla riduzione del debito pubblico. Non avevo detto prima nell'intervento che, per quanto riguarda le risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalla manovra di bilancio, le stesse saranno assicurate dai seguenti ambiti di intervento: la rimodulazione di alcuni fondi di investimento e l'avvio di un programma di revisione e riqualificazione della spesa della pubblica amministrazione; la revisione di alcuni sussidi dannosi dal punto di vista ambientale; incrementi di gettito derivanti dal miglioramento della *compliance*, correlati anche all'incentivazione all'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento; gettito addizionale derivante dalla crescita generata dal programma di investimenti (tale retroazione fiscale è inclusa, parzialmente, nelle stime solo a partire dal 2022);

pur con le note difficoltà di rapporto con tali categorie, è bene ricordare che, per la prima volta nella storia, essi sono stati considerati dallo Stato quando c'era da fornire supporto finanziario. Non era mai successo prima che ricevessero qualcosa. Mi riferisco al fondo di ultima istanza del decreto cura Italia, con il contributo anticipato delle casse per questioni di rapidità, ma in realtà erogato dallo Stato. Se ho capito bene, il collega De Bertoldi ha detto che la logica del Governo è, o è stata in passato, colpire i ricchi. Ma in questa fase pandemica, nella quale si è trovato a dover fronteggiare una situazione catastrofica mai avvenuta prima, l'intenzione del Governo è stata, *in primis*, quella di tutelare le fasce deboli della Nazione. Allo stesso tempo, si è cercato di dare un supporto alla fascia produttiva del Paese, ma mai si è avuta alcuna intenzione di colpire qualcuno. Di certo, non si è portata a termine - come diceva correttamente la senatrice Rauti - la legge delega sulla riforma fiscale, alla quale, comunque, il Governo sta lavorando, perché non c'era spazio, *in primis* temporale e in secondo luogo economico, per poter agire. Come sapete, infatti, qualsiasi ipotesi di riforma fiscale che possa abbassare in maniera sensibile il livello di tassazione deve essere ponderata e passare anche per la correttura di bilancio; e di certo non si può fare una riforma in uno stato di emergenza. E nel 2020 avevamo e abbiamo soltanto da lavorare per far ripartire il Paese. L'intenzione del Governo, di qualsiasi Governo, è fare una riforma fiscale. Saremmo meschini se addebitassimo a qualsiasi Governo in carica in questa fase, in questo 2020, il fatto di non aver portato a casa questo progetto. È stato detto che abbiamo salvato le banche. A parte il fatto che con l'espressione «salvare le banche», in realtà, si dovrebbe intendere non salvare i banchieri, ma salvare il tessuto produttivo che sta intorno alle banche; quelle imprese che hanno richiesto affidamenti perché ne hanno bisogno per lavorare e far continuare a lavorare e vivere i loro dipendenti, i banchieri che hanno le loro responsabilità per aver portato le banche in quelle condizioni risponderanno delle loro azioni. Deve, però, pensarci la magistratura, e non noi. Ricordo che noi siamo la parte legislativa di questo sistema. E ricordo - solo per dire quanto questa cosa sia vera - che, mentre il Governo ha salvato recentemente la Banca popolare di Bari, contemporaneamente la magistratura sta istruendo i processi nei confronti dei dirigenti che hanno distrutto quella banca. Apprezzo con piacere quanto detto dal senatore Monti in merito alla definizione del *recovery fund* come migliore strumento e maggiore fonte di preoccupazione allo stesso tempo. Questo ci deve portare a capire che l'utilizzo che ne faremo e il sostegno che daremo a questo Governo - ciascuno per la propria parte, le forze politiche presenti in Parlamento - saranno fondamentali per lavorare al meglio, e non solo per non sprecare la pioggia di miliardi che arriverà, ma anche per utilizzarla in maniera efficace ed efficiente, che sia la nostra ultima possibilità di recupero. Siccome partiamo da un livello di debito superiore rispetto agli altri Paesi, dobbiamo sfruttare al massimo questa possibilità, non sprecando neanche un centesimo.

Ricordo che, quando un paio di anni fa venne a trovarci l'assessore ai lavori pubblici di Bilbao e venne a sapere il costo delle nostre rotonde, ci fece presente che da loro, a Bilbao, costavano circa quattro volte di meno, confermando quei livelli di costo. Ciò vuol dire che sia ai livelli alti che a quelli bassi ci sono problemi del genere che vanno risolti.

perché non c'è mai limite al peggio, ma non per questo si deve andare a ipotizzare la catastrofe in uno scenario, altrimenti non basteranno tutti i soldi del mondo. Quindi, la migliore delle cose da fare è ipotizzare sì uno scenario peggiorativo, ma con un livello di probabilità estrema; non si può considerare tutto. Concordo però con una cosa: c'è bisogno di tutti e proprio per questo dobbiamo tutti cominciare a fornire supporto al Paese, partendo dal nostro piccolo qui in Senato. Se vogliamo che i nostri e i vostri provvedimenti siano accettati, allora cominciamo a lavorare insieme qui dentro, indipendentemente dal Governo.

cerchiamo di combatterci politicamente sui dati di fatto e non utilizziamo il nostro tempo e il nostro fiato per smontare le *fake news*. Ricorderete che ieri il presidente Perilli ha dovuto riorganizzare il suo intervento per rispondere alle false notizie date dal senatore Salvini. È stato

livelli pre-Covid. Se vogliamo essere precisi - ora devo dare dei numeri, cosa che non mi piace fare - dopo i ribassi del secondo trimestre (-18 per cento l'elettricità e -13,5 per cento il gas), continuati anche nel terzo trimestre, con il rafforzamento della ripresa delle attività economiche è arrivato un rimbalzo dei prezzi dell'energia. Ma per quanto riguarda gli effetti sui consumatori, nel 2020 la famiglia tipo beneficerà comunque di un risparmio complessivo di circa 207 euro rispetto al 2019. Nel dettaglio,

- come diceva il senatore Paragone - ma non dobbiamo andare a dire in giro cose non corrette. È opportuno aprire il mercato dei servizi a una maggiore offerta; in questa maniera i cittadini avranno notevoli benefici diretti.

ma non mi pare che per anni la destra abbia fatto qualcosa in merito, anzi. Invece, la legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia; nel 2021 verranno trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità, il cosiddetto *bonus* bebè, e il *bonus* asilo nido e ulteriori risorse saranno indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché di riordino e sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Persino nel corso dell'emergenza Covid sono state incrementate le risorse dei fondi sociali per la non autosufficienza, Dopo di noi, Fondo politiche della famiglia) con la finalità di rafforzare il sistema degli interventi dei sistemi territoriali dedicati alla famiglia e alla disabilità. Possiamo giustamente avere posizioni politicamente diverse, ma ritengo corretto riportare quello che è stato fatto in questo periodo dal Governo; si tratta di attività che - ripeto - nessuno avrebbe mai pensato di dover gestire in così poco tempo e per le quali il supporto di tutti, anche in questa fase di approvazione dello scostamento

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il verificarsi di una situazione inedita come quella causata dal Covid-19 ha sicuramente provocato scenari economici di difficile previsione. Siamo anche consapevoli che l'ottimismo è una componente fondamentale per cercare di superare al meglio le difficoltà, ma quell'ottimismo non deve trasformarsi in una mancanza di presa di coscienza di quelli che potranno essere gli scenari futuri. La sensazione è che stiamo drammatizzando la situazione sanitaria, provocando paure forse eccessive - mi ricollego al discorso della senatrice Rivolta - e sdrammatizziamo la situazione economica, facendo previsioni troppo rosee sugli indici economici per il 2020 e per i prossimi anni.

L'Ufficio parlamentare di bilancio è quindi il primo a mettere in guardia su queste stime. Inoltre, la NADEF prevede un aumento del 4 per cento dei contributi sociali nel triennio 2021-2023, ma sconta la mancata stima dell'impatto della decadenza del divieto dei licenziamenti al 31 dicembre 2020, in termini di

ma il problema resta ideologico. Siamo tutti consapevoli delle problematiche e spesso nell'individuarle diciamo le stesse cose: bisogna agire con velocità;

non lo nego assolutamente, ma oggi siamo in emergenza economica e c'è bisogno di una spinta seria sul PIL. Il rapporto debito-PIL si attesterà al 158 per cento, ma oggi il Fondo monetario internazionale fa invece una stima del 161 Allora bisogna far risalire il PIL, quindi il denominatore del rapporto. Purtroppo, il PIL è un numero ci vuole concretezza: bisogna mettere in moto l'economia. la crescita del PIL si crea dando slancio all'economia reale; l'occupazione si crea se ci sono le aziende che danno lavoro. È una ricetta da noi proposta, ma questa maggioranza sembra essere sorda ad uno *shock* fiscale. La pressione fiscale nel 2020 è prevista collocarsi al 42,5 per cento e al 42,6 per cento negli anni successivi: questi sono i dati della NADEF. Ma in realtà la pressione fiscale sulle società è tra le più elevate in Europa:

calcola che in realtà la pressione fiscale, depurata dal sommerso, arriva a superare il 48 per cento. Le aziende hanno bisogno non di tanti sussidi, ma di non essere tartassate; hanno bisogno di meno burocrazia. Vi rendete conto che le grandi aziende - quando ancora producono in Italia - ma dichiarano i profitti in altri Paesi europei? Vogliamo far rimanere i profitti in Italia? Allora ci deve essere una competitività anche nella tassazione e la competitività dell'Italia si misura anche sulla velocità degli interventi. Tutti i disegni di legge collegati quando vedranno la luce? Quando avranno ricadute reali sui cittadini italiani? Annotati su questa NADEF ci sono tanti disegni di legge e tante belle parole, ma le parole non bastano più: devono tramutarsi in provvedimenti che abbiano effettivamente un impatto strutturale e a lungo termine termine sull'economia nazionale. Quindi, ci vogliono una profonda revisione del sistema fiscale che riduca la pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese *(Applausi)*; una semplificazione una sburocratizzazione vera; inoltre, investimenti strutturali che vadano dalle opere pubbliche al potenziamento dell'istruzione e della ricerca. Abbiamo fatto 100 miliardi di debito e ne abbiamo 84 fermi in cassa: questo è indice di quanto sia macchinoso e complesso il meccanismo. Questi soldi li vogliamo spendere? Noi abbiamo le ricette: medicina territoriale, medici di base, telemedicina, investimenti sull'edilizia sanitaria, sostegno dell'*automotive*, turismo, ristorazione e commercio, tassazione aziendale. Ascoltateci: noi le ricette concrete le abbiamo.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

economia e finanza ha il merito di cercare un equilibrio tra prospettive di breve e di lungo termine, ponendo le politiche espansive in relazione alla sostenibilità del debito attraverso un percorso costante di riduzione del *deficit* nominale e del rapporto debito-PIL; un tema di cui non si parla molto, ma che invece è di importanza fondamentale per un Paese che non potrà contare per sempre sull'attivismo della BCE sui mercati. È anche una questione di carattere morale verso le future generazioni, alle quali va lasciata un'economia non schiacciata dal macigno di un debito ancora più grande di quello che noi abbiamo ereditato. Allo stesso tempo è apprezzabile che le stime vengano fatte seguendo un principio prudenziale, senza, cioè, tenere in considerazione l'effetto delle riforme in cantiere. Pur tuttavia, la bontà di tali previsioni si scontra oggi con una grande incognita, che si chiama andamento della pandemia. Non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane in Italia, in casa nostra; ma non sappiamo neanche cosa succederà a livello internazionale, e soprattutto quali saranno le misure restrittive che verranno prese nel mondo per contrastare la diffusione del virus. Non è una questione di poco conto per tutti quei settori economici che prima del Covid avevano la principale fonte di redditività nelle esportazioni; un grande punto di domanda a cui nessuno può fornire oggi delle risposte, se non attraverso maggior raccordo sulle politiche di prevenzione a livello europeo. Quello che invece dobbiamo puntare a governare è l'andamento del mercato interno, partendo dal presupposto che politiche per contrastare la diffusione del virus e politiche per il rilancio economico di questo Paese sono il rilancio economico di questo Paese sono due facce della stessa medaglia. Per questo, più che di nuove restrizioni, abbiamo bisogno di maggiori controlli, di fare continui appelli al senso civico, spiegando sempre che le sorti delle persone più fragili, dei nostri anziani, delle imprese, dei posti di lavoro passano dal comportamento di ciascuno di noi.

bar, attività di ristorazione con le chiusure anticipate, e a tutto l'indotto dello sport dilettantistico, è fortemente danneggiata. A ciò si sommano i problemi del turismo, della cultura, del commercio al dettaglio: quei settori che, fino a quando non sarà sconfitto il coronavirus, vivranno sulla soglia di galleggiamento. Per questo dobbiamo archiviare la stagione del cura Italia, l'ora giusta degli aiuti a pioggia, perché allora non si capiva ancora come si sarebbero

e concentrarci su quei settori che, da gennaio, possono far esplodere la questione occupazionale. È una delle più grandi preoccupazioni a livello economico, la questione occupazionale, una volta terminati gli interventi su cassa integrazione e ammortizzatori sociali fin qui Dobbiamo agire con la consapevolezza che qui è in gioco la coesione sociale. Quello che voglio dire è che, nella legge di bilancio, lo sforzo di prospettiva non deve far perdere di vista le necessità immediate e concrete, riflettendo in questo lo schema e lo spirito della Nota di aggiornamento in esame, in cui breve e lungo termine, visione e concretezza hanno la stessa attenzione e importanza. È un punto dirimente, come lo è quello sulla crescita, a cominciare dalla riduzione del costo del lavoro, per rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie, e dalla riforma del fisco, che generi una maggiore equità sociale, per poi arrivare alla crescita alimentata dall'aumento degli investimenti, pubblici e privati, anche in conseguenza degli ingenti mezzi che ci perverranno dall'Unione europea. Se però davvero vogliamo che l'Italia produca una crescita in grado di rafforzare il rimbalzo del PIL nei prossimi due anni, dobbiamo vincere soprattutto una partita: quella contro la burocrazia, per migliorare efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. Solo con una pubblica amministrazione attrezzata, preparata e veloce sarà possibile avviare tutti quegli investimenti necessari per garantire la crescita auspicata, ma anche indispensabile. Come ha ricordato il ministro Gualtieri in Commissione, serve un miglioramento della capacità di spesa e di programmazione della pubblica amministrazione, ma anche un costante sfoltimento delle norme e delle procedure e un nuovo patto col sistema bancario, per scongiurare una prematura stretta al credito. Occorre intervenire velocemente su questi elementi di sistema, andare avanti col percorso intrapreso con il decreto semplificazioni, superare agilmente le criticità che stanno emergendo sull'applicazione delle misure pilastro, come quella che riguarda il superbonus al 110 per cento. Serve però anche un terzo elemento, che faccia da anello di congiunzione tra fisco e pubblica amministrazione, ossia la riforma della giustizia, che - come sappiamo tutti - costa ogni anno all'Italia un punto di PIL e costituisce il principale elemento ostativo agli investimenti stranieri, di cui abbiamo forte bisogno. Riforme radicali in questi settori sarebbero il più grande moltiplicatore economico che il Paese abbia mai visto, per darci una base forte, in grado di reggere l'urto della pandemia, e soprattutto in grado di raggiungere quegli obiettivi di crescita e di sostenibilità del debito, di cui parlavo in precedenza. Anche per questo serve, nei prossimi mesi, un grande investimento sui giovani del Paese. I giovani sono uno straordinario giacimento di competenze, di energie e di visioni innovative, che devono essere liberate. Sono loro che soffrono di più in questa pandemia e lo vediamo anche guardando ai numeri del mercato del lavoro. Anche se fino adesso ha tenuto, vediamo che la disoccupazione giovanile sta aumentando. I giovani devono essere messi al centro del processo per la modernizzazione di un sistema, che

ribadendo quello che abbiamo detto ieri sul *recovery fund*: sappiamo che la strada non sarà per niente semplice, che ci saranno delle difficoltà e che la riuscita dell'operazione passa dalle riforme di sistema che richiedono grande coraggio e grande decisione, ma la strada intrapresa dal Governo è quella giusta. Per queste ragioni, voteremo a favore della Nota di aggiornamento ed esprimeremo un voto favorevole alla risoluzione presentata dalla maggioranza.

Quindi, mi ripasso l'intervento e ascolto le singole lagnanze su tutto quello che nel Paese non va. Devo dire che è bravo, Presidente, perché non ne dimentica una, tutto l'intervento è stato fatto elencandole tutte, un po' come il *cahier de doléances* della Rivoluzione francese, contenente tutte le lamentele che venivano rivolte al Parlamento prima della Rivoluzione; anche un po' come una sorta di "Onda Verde" sul traffico e quindi su tutte le criticità degli spostamenti e delle automobili. Dalla camicia verde è passato Accanto a lui, che è ormai l'Al Bano della politica italiana, c'è la Romina, che è la Meloni: anche lei ogni mattina ci diletta con i suoi comunicati stampa nell'elenco delle lagnanze e delle cose che non vanno. Stamattina ho letto il comunicato in cui veniva indicato il tema vero dei ristoratori che sono penalizzati da questa crisi dei bar, delle palestre e delle attività sportive, che tra l'altro con la chiusura dovuta dovuta al coronavirus e con la stagione invernale alle porte, quindi con maggiori difficoltà, avranno sicuramente bisogno di altro sostegno da parte dello Stato; c'è poi l'industria del matrimonio e del *catering*; le gite scolastiche; le agenzie di viaggio e gli alberghi in genere. È un un lungo elenco che credo in quest'Aula nessuno possa dire di non condividere, perché oggettivamente, a seguito della pandemia, ci sono alcuni settori e alcune categorie dell'economia del nostro Paese che stanno risentendo più pesantemente della crisi ed è quindi necessario intervenire. Poi naturalmente Salvini ci ha ricordato anche gli alluvionati del Nord-Ovest, su cui vi

con una sorta di dichiarazione nei confronti del Presidente del Consiglio di un amore mancato e non ricambiato: «telefonami, perché se tu mi telefonassi, probabilmente potrei risponderti e potrei anche darti dei suggerimenti su cosa fare». Ha detto che ascoltano. Quando viene a mancare il filo del dialogo fra la maggioranza e l'opposizione, stare lì a cercare il responsabile mi sembrerebbe un po' un errore, perché magari le responsabilità sono reciproche, però so una cosa, Presidente: rispetto

dovremmo avere la forza, se proprio non riusciamo a trovare l'unità nei contenuti, di trasformare in una sorta di voto tecnico. Mi riferisco allo scostamento, su cui c'è la necessità di una maggioranza qualificata. Non c'è una maggioranza che è senza i numeri, e lo dimostreremo anche oggi, ma c'è una condizione oggettiva di difficoltà legata ad una pandemia che ha colpito anche dei colleghi. Noi abbiamo dovuto fare i salti mortali per far sì che tutti fossero presenti e credo che questa occasione (è un ulteriore appello che faccio a tutte le forze dell'opposizione) e questa condizione particolare potrebbe spingere il Parlamento a tracciare il primo segnale di unità e di collaborazione. Ciò non vuol dire far parte della maggioranza, non vuol dire condividere responsabilità, ma vuol dire soltanto che di fronte ad una divisione che c'è nel Paese, si fanno però prevalere le necessità dell'Italia e del Parlamento di riuscire a trovare numeri su una maggioranza qualificata che altrimenti rischierebbe di venir meno. Per cui l'appello che faccio è: non limitatevi all'elenco delle cose che non vanno, ma partecipate insieme a noi al voto sulla risoluzione, perché caro Salvini e cara Meloni, se non ci fosse la maggioranza che qui si organizza con i senatori fatti venire anche febbricitanti, con tamponi negativi (ci tengo a sottolinearlo), tutto tutto quell'elenco delle cose che ci avete raccontato non troverebbe soluzione, perché non ci sarebbero le risorse economiche per sostenere tutte quelle categorie che ci hanno detto essere in difficoltà. Per cui l'appello ulteriore che faccio all'opposizione è, almeno almeno sullo scostamento, di votare insieme; poi sulla NADEF, che è il provvedimento politico per eccellenza, ci divideremo un'altra volta. Ma io credo che questo appello debba essere raccolto, così come credo che

Oggi abbiamo letto anche di Giorgetti che parlava di populisti e popolari che diventano popolaristi, con salti diciamo dialettici che comunque

ex amici di Bagnai che sono guidati da Orban sostanzialmente sul tema dei diritti che devono essere legati ai finanziamenti. Davanti a tutte queste sfide credo vi sia la necessità di avere un'Italia forte

condizione di difficoltà e di debolezza, diventando quasi una Nazione obiettivo. Per evitare tutto questo abbiamo il dovere, Presidente, di utilizzare quelle risorse al meglio, perché bisogna uscire celermente da questa condizione di difficoltà anche rispetto agli altri Paesi europei che sono più forti. Quindi è decisivo capire non solo come spendere le risorse, ma soprattutto come investirle. Abbiamo il dovere di sostenere i progetti più importanti e di accompagnarli oltre che con risorse economiche anche con riforme strutturali. Si è fatto riferimento alla riforma della giustizia e alla sburocratizzazione, tutte riforme necessarie affinché quelle risorse si spendano e si spendano bene. Altre risorse devono essere destinate alle politiche attive per il lavoro. Per una fase abbiamo sostenuto sostenuto esclusivamente quelle passive come la cassa integrazione, abbiamo impedito la disoccupazione e la possibilità di licenziare, giustamente. Il problema è che ora la fase è cambiata. è cambiata. Quando scopriremo il vaccino, non migliorerà la situazione economica. Quando avremo scoperto il vaccino, non potremo non potremo dire che il Paese sarà uscito dall'emergenza economica, anzi, sarà una fase ancora più complicata e delicata, dunque bisogna intervenire in questa direzione per creare lavoro. Bisogna sostenere le imprese sulla formazione e sull'innovazione perché la nostra economia cambierà. Bisogna accompagnare le imprese ad una conversione occupazionale e di *mission*, così come bisognerà intervenire sulle infrastrutture, il Ponte o qualunque collegamento che resti, che ritengo siano indispensabili per creare ricchezza. Dobbiamo pensare che investiamo 54 miliardi di euro in tre anni per reddito cittadinanza e quota 100, mentre il Ponte costa 4 miliardi, ma crea ricchezza che resta perché dà al nostro Paese una centralità che costruisce ulteriore economia. Ci rendiamo conto, quale è la spesa produttiva e di quale rischia di essere una spesa di assistenza che non genera ricchezza futura. Concludo dicendo che bisognerà sostenere, come penso il Governo farà, i più fragili e i più penalizzati da questa pandemia, che sono le persone con disabilità, gli anziani e anche gli studenti che hanno avuto difficoltà nella formazione e dico, infine, che dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che vengono messi a disposizione. L'idea che l'Italia si rassegni a prendere 5 miliardi di euro, che sono le risorse che perderemmo in dieci anni non utilizzando il MES, non riesco a tollerarla. Con 5 miliardi di euro in questo Paese si potrebbe fare tanto: eliminare le file per i tamponi, eliminare il fatto che ci siano medici di base che dicono che hanno disponibili 30 vaccini con 300 richieste; potremmo intervenire sulle specializzazioni mediche. Perché questi 5 miliardi di risparmio che potremmo avere...

perché crede nelle politiche espansive messe in atto dall'Unione europea e perché sappiamo che questo Paese sarà nelle condizioni di utilizzare al meglio queste risorse, soprattutto per dare una mano alle nuove generazioni, che sono quelle che ce le stanno prestando.

descrivendo la situazione certamente difficile che stanno attraversando il nostro Paese e la nostra economia ed evidenziando chiaramente come le misure messe in campo dal Governo, potenza di fuoco secondo il nostro Presidente del Consiglio, si siano rivelate insufficienti.

di medio e lungo periodo per quanto riguarda lo sviluppo del Paese. È evidente che questa volta con questa Nota abbiamo un vantaggio rispetto agli anni precedenti: grazie alla

maggiore serenità per quanto riguarda l'approccio alla legge di bilancio, che è *in itinere* e di cui, tra qualche giorno, si inizierà a parlare, ma noi mettiamo sempre al centro del nostro volere politico ciò che abbiamo sempre detto e, cioè, che è stato giusto tutelare e risarcire i redditi e l'occupazione perché in questa fase serviva anche questo,

alcuni interventi anche di colleghi di maggioranza. Il senatore Pittella ha fatto riferimento al ritorno del Patto di stabilità e, quindi, era in qualche modo molto preoccupato. Senatore, condividiamo questa sua preoccupazione. A tale riguardo, infatti, diciamo che sarà necessario un ritorno graduale a questo sistema: bisogna ritardarlo, perché addirittura l'Europa già pensa che con la prossima primavera o con la prossima estate si possa tornare alla rigidità che c'è sempre stata. non sarà possibile evidentemente, perché in un contesto di incertezza, con una ripresa così disomogenea, come ci hanno detto anche i rappresentanti del Governo che si sono succeduti in questa discussione, non si possono minare tutti gli sforzi che in questi mesi sono stati

che ancora aspettano di vedere la luce dopo l'approvazione dei decreti riferiti al post-Covid. Ci sono poi cose anche abbastanza bizzarre in questa Nota di aggiornamento. Voglio ricordare l'introduzione del salario minimo, fine certamente nobile, ma, prima di chiederlo ai datori di lavoro privati, che stanno in qualche modo soffrendo rispetto all'emergenza sanitaria c'è stata, iniziate ad adeguare gli stipendi dei dipendenti pubblici, in particolare delle Forze dell'ordine e degli insegnanti, che percepiscono paghe ridicole dallo Stato che, in questo caso, è il loro datore di lavoro. Non voglio parlare poi della delega alla riforma fiscale. Lo scorso anno annunciavate

mai come ora nella storia del Paese ci sarebbe bisogno di un Governo stabile, capace di guidare i processi di sviluppo dell'Italia. Come ho detto, questo è un libro dei sogni, una sequenza di numeri che alzano le previsioni positive e, quando serve, abbassano quelle negative. Che dire poi dei fondi del *recovery plan*? Come pensate che qualcuno possa credere che voi abbiate la capacità di spendere queste risorse in una visione di insieme, dopo che avete utilizzato 100 miliardi

Ad oggi non riusciamo a vedere un effetto tangibile di quanto vi vantate di avere fatto per il Paese. La tanto annunciata potenza di fuoco, di cui ha parlato il presidente Conte nei mesi scorsi, si è ridotta ad una candela consumata, tra l'altro anche molto velocemente. comunque stati bravi e capaci di impartire ordini. Dite agli italiani che devono fare attività motoria con le mascherine e che possono correre anche senza; possono andare ai matrimoni con 30 invitati e indicate perfino quante persone possono entrare nelle nostre abitazioni private. Siete capaci di scatenare contro gli italiani i droni, gli elicotteri, chiamando anche i vicini di casa nostra a fare da delatori. Guai a non rispettare le distanze, a non rispettare le regole, ma poi consentite tutti i giorni a decine di imbarcazioni

a strappare oggi l'approvazione del documento, dovete accettare la verità dei fatti di non avere più la forza di andare avanti, né il sostegno del Paese, che non ha mai votato che non ha mai votato questa coalizione innaturale, nata solo per ostacolare il centrodestra, che è la vera maggioranza di questo Paese. Provate pure a fare appello, come ho sentito fare oggi dal collega Paragone e da tanti altri colleghi, senso di responsabilità che chiedete a noi ma che voi mai avete dimostrato in tutti questi mesi, con la bocciatura di tutte le proposte che i nostri *leader* e i Gruppi parlamentari hanno presentato. Sicuramente potrete far breccia su qualcuno per raggranellare qualche voto sparso qua e là, ma state certi che non potrete contare su Fratelli d'Italia perché noi non daremo mai un voto e il sostegno a questo Governo.

di risoluzione presentate dalla maggioranza. La NADEF evidenzia in modo eclatante la straordinarietà della fase: 100 miliardi di euro di indebitamento e la gestione dell'emergenza. Colleghi, ho ascoltato con attenzione il dibattito e devo dire che,

Vorrei provare a proporvi una lettura che ci consenta di riconoscerci

cassa integrazione e agli interventi straordinari (non ancora pienamente soddisfatti per la cassa integrazione). Guardate che l'obiettivo primario - vorrei che su questo

o di evitare che all'emergenza sanitaria drammatica si saldasse un'emergenza sociale fuori controllo. Da questo punto di vista, colleghi e colleghe,

È un dato oggettivo e non capisco perché dobbiamo insistere, certamente per il posizionamento politico, ma mi chiedo a cosa serva. Venendo al secondo molti colleghi ci hanno detto che la Nota di aggiornamento è il libro dei sogni, che le previsioni sono aleatorie, aleatorie, ma c'è qualcuno nel mondo che sia in grado di fare previsioni certe su quello che accadrà nei prossimi tre anni in questo mondo, nell'intero pianeta? C'è qualcuno qui che è in grado di alzarsi e di dirlo? Non c'è organismo internazionale che non metta al centro del ragionamento il tema della pandemia e dei rischi che la ripresa della pandemia propone sull'economia. Vorrei anche ricordare che perfino il Fondo monetario internazionale ha detto che le esperienze che ci stanno alle spalle sui *lockdown* non hanno prodotto un danno all'economia,

che non va sottovalutata. Non ho mai usato aggettivi superlativi in relazione alla gestione del Covid e continuo ad evitarlo. Sono preoccupato perché c'è una novità in Italia che riguarda la diffusione in tutto il Paese del Covid, con caratteristiche del sistema sanitario oggettivamente diverse. Del resto, sono anni che parliamo delle distanze anche abissali tra il Servizio sanitario del Nord e quello del Sud.

Questo è il vero problema. Forse mi viene da dire, per fare una provocazione, che sarà il caso di pensare a delle case della salute temporanee per prendere in carico nel territorio al Nord e al Sud

Dunque, il richiamo a lavorare insieme, dunque, non è una richiesta di corresponsabilità, come ho sentito dire ieri in relazione magari alla preoccupazione che non si raggiungano gli obiettivi che ci stiamo proponendo. No.

La manifattura ha reagito meglio, molto meglio. I nostri problemi, in primo luogo, sono sui servizi. In primo luogo sul turismo, sulla ristorazione sul sul commercio, sulle fiere, su questi servizi dobbiamo continuare a fare interventi di emergenza. Lo chiamate assistenzialismo? No. Essi sono mirati a tenere aperte le imprese, a tenerle in piedi e a costruire un ponte in un processo di cambiamento. Dunque, da una parte, dovremo continuare queste politiche e, dall'altra, fare quel salto di qualità che è indispensabile. Discutiamo, allora, di questo salto di qualità. Noi dobbiamo cominciare, con il bilancio, a investire strategicamente, con le risorse del *recovery le risorse del *recovery fund*, sull'avvio di un processo per un nuovo modello di sviluppo e un nuovo modello sociale. Dobbiamo investire sulle periferie, le diverse periferie, territoriali e sociali, sul Sud in primo luogo, ma anche sulle aree interne. E dobbiamo investire sul Sud e sulle aree interne, in primo luogo per disegnare quel nuovo modello di sviluppo, quella transizione ecologica dell'economia. Ma questa, colleghi, è una sfida che possiamo portare avanti insieme anche laddove non riconoscessimo la stessa identica impostazione sulle risoluzioni. Qualcuno ha ricordato il Piano Marshall, Togliatti, De Gasperi, Nenni, quella fase storica. Guardate che ci trovavamo trovavamo nel più duro scontro ideologico. Nessuno risparmiava nessuno. C'era chi mangiava i bambini e c'era chi denunciava chi mangiava i bambini, ma c'era la capacità di vedere avanti e di trovarsi su alcuni punti di fondo. Questa è la politica. La politica non è l'elenco di ciò che non va. La politica non è distruggere ciò che c'è. La politica è costruire il progetto, almeno mettersi insieme per un pezzo di strada. Non vi chiediamo corresponsabilità. Vi chiediamo di provarci, sapendo quant'è difficile, dovendo fare le riforme, dure e impegnative: quella fiscale, quella della pubblica amministrazione. O facciamo questo passo,

il voto di oggi sullo scostamento di bilancio e sul NADEF quest'anno, davvero e al di là di ogni retorica, come abbiamo sentito nella discussione, rivestono un'importanza straordinaria, decisiva, per il Paese, per gli italiani e per il loro futuro. Noi dobbiamo far fronte, come i dati di oggi sembrano confermare, alla pesantissima crisi provocata dalla pandemia; occuparci e farci carico dei suoi effetti sulla vita concreta delle persone, delle famiglie e delle imprese. Allo stesso tempo dobbiamo investire sulla ripresa e progettare il futuro, avviando una stagione di riforme necessarie non solo per superare i problemi prodotti dall'emergenza pandemica,

è possibile, perché per affrontare questa sfida il Paese ha l'opportunità storica di poter contare sugli strumenti straordinari che l'Europa sta mettendo in campo, come il *recovery fund*, o che ha già messo in campo, come le risorse destinate alla ricerca o ad affrontare la disoccupazione finanziando gli ammortizzatori sociali. Risorse per cui questo Governo si è battuto in Europa e che abbiamo ottenuto con uno sforzo collettivo di tanti Paesi e di tante forze che sono tornate a credere nell'Europa. Si tratta di tante risorse; lo voglio dire senza fare una battuta, ma seriamente. ma seriamente. Io credo che sia positivo che chi quelle risorse non le voleva oggi voglia contribuire a spenderle, nell'interesse del Paese. Ma l'utilizzo delle ingenti risorse di cui abbiamo parlato, anche ieri, non può non essere accompagnato da riforme decisive e ineludibili, prima di tutto quella fiscale; una riforma che deve essere equa, ridurre il prelievo e proseguire sulla strada che questo Governo ha intrapreso con il taglio del cuneo fiscale e la riduzione della tassazione per i lavoratori dipendenti. Serve rafforzare la lotta all'evasione fiscale, che non è un accanimento o una fissazione di una sinistra statalista, ma che oggi è necessaria. Oggi i dati dell'Istat ci dicono che il

radicale della pubblica amministrazione, anche accelerando le norme sulla digitalizzazione previste nel decreto semplificazione e aprendola ai giovani. Riforme quindi dall'altra, il tema delle infrastrutture, del digitale, di reti che accelerino e velocizzino la mobilità. Penso che con questa Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza ci siano le condizioni per rispondere alle tre priorità che non solo il Governo, ma il Paese intero devono affrontare. Prima di tutto abbiamo tutti il dovere di aiutare le persone e le imprese più colpite dalla crisi pandemica. Il dovere delle istituzioni tutte oggi quello di proteggere chi è in difficoltà e di non lasciare nessuno da solo. Servono le risorse per non interrompere, anche uscendo da una logica emergenziale, il sostegno - è grave che qui qualcuno l'abbia definito sperpero - che in questi mesi è stato comunque garantito a tanti, se non a tutti, di fronte alle difficoltà. Serve riformare gli ammortizzatori sociali e il sistema di protezione sociale, per garantire un aiuto a chi non l'ha mai avuto. Fino alle iniziative - non dimentichiamocelo - non dimentichiamocelo - assunte dal Governo per rispondere alla pandemia: lavoratori autonomi, partite IVA, lavoratori delle piccole imprese non sono mai ora diciamo che non vanno mai più lasciati soli di fronte alle difficoltà, come non sono stati lasciati soli in questi mesi difficili. Serve anche attenzione per continuare a sostenere le imprese, quelle che soffrono di più, quelle dei settori che sono stati più esposti alla crisi. Aiutare le persone oggi significa anche investire sulla sanità, sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini; dobbiamo continuare a farlo, investendo, come dice la NADEF, tutte le risorse necessarie. Il secondo obiettivo prioritario è quello di rilanciare l'economia. Servono misure anticicliche come il *bonus* del 110 per cento, che dovrà essere prorogato oltre la scadenza oggi prevista; servono politiche di coesione territoriale, ma serve soprattutto investire scegliendo una strada. Nella NADEF la scelta c'è: è quella dello sviluppo sostenibile, della *green economy,* della digitalizzazione e della valorizzazione dei talenti di questo Paese, quelli artistici, naturali e delle donne, del cui

Il terzo obiettivo, anzi, la terza priorità è forse la meno scontata, ma anche la più necessaria, quella che deve sempre restare nel *target* di ogni politica che faremo da oggi in avanti. Il punto è che serve un'idea di futuro, sapendo che sbaglia chi pensa o addirittura auspica che il post-Covid ristabilisca o possa ristabilire le condizioni pre-Covid. Non sarà così. In realtà avremo di fronte una transizione dagli esiti non scontati. Questi mesi di pandemia cambieranno, anzi hanno già cambiato il modo di lavorare. Lo *smart working* spingerà le imprese a riorganizzarsi, la mobilità cambierà; probabilmente cambieranno o stanno già cambiando i tempi e le abitudini di vita, i comportamenti delle persone; le nostre città cambieranno, i centri dedicati ai servizi per i lavoratori degli uffici non reggeranno più come li abbiamo conosciuti. Abbiamo di fronte una transizione che o si subisce o si governa per migliorare la vita delle persone, per farne un'occasione, un'opportunità di vita e di lavoro. Questo è il compito della politica e delle istituzioni, non solo del Governo. Abbiamo di fronte la sfida di saper guardare alla realtà e immaginare e realizzare un futuro migliore per il Paese, il Paese, in un'Europa che si è riscoperta forte, ha riacquistato il senso di sé e, per molti versi, ha ripreso la strada che i suoi fondatori avevano pensato. È una sfida talmente grande, quella che abbiamo di fronte, che davvero le polemiche sterili e i tentativi di ridurre tutto a un teatrino tra maggioranza e opposizioni sono stucchevoli. Per questo, anche la non serve al Governo o alla maggioranza, ma al Paese e ai cittadini. Anche le ultime elezioni hanno dato un messaggio chiaro: i cittadini chiedono serietà, affidabilità e responsabilità; hanno premiato tutti i candidati uscenti, per questo. Non c'è la rendita di posizione garantita per chi sa solo agitare i problemi. Oggi, di fronte alla crisi, si chiedono risposte concrete alla politica e alle istituzioni.

rappresentanti del Governo, colleghi senatori, a sei mesi dall'approvazione del Documento di economia e finanza,

sono e qual è la situazione attuale. Abbiamo dati cristallizzati, sui quali oggi costruire una proposta presente e futura per il rilancio del nostro Paese.

Paese. Sicuramente l'insuccesso dei vostri provvedimenti è dovuto alla frammentazione: ne avete fatti troppi sin dal primo giorno. Le opposizioni e Forza Italia vi hanno proposto uno scostamento unico di 100 miliardi di euro *(Applausi)* per scrivere

Soprattutto negli ultimi giorni e nelle ultime ore, in un momento così particolare, in cui gli italiani si aspettano provvedimenti a loro favore, cosa fa il Governo (o meglio, meglio, una sua parte)? Nomina come presidente di Unicredit un esponente del Partito Democratico della banca più importante. *(Applausi)*. Invece di pensare agli italiani, si pensa a occupare le banche. E tutto questo passa

che non sono mai partiti, come il *bonus* mobilità o il *bonus* vacanze, che sono stati assolutamente inutili e hanno sortito un effetto assolutamente contrario. A fronte di queste misure, poco o niente si è fatto invece per gli investimenti, che sono il vero volano e il vero moltiplicatore dell'economia. Dalla NADEF e dai dati - leggiamoli, che sono inconfutabili - possiamo dire che la parte degli investimenti,

troppo poco per pensare al rilancio del Paese e alla ripartenza dell'Italia. *(Applausi)*. Basate invece questa relazione tutta su previsioni ottimistiche, costruite assolutamente sulla sabbia, e si capisce chiaro e tondo che le guardate anche con la chiave di lettura elettorale del prossimo 2023. *(Applausi)*. Anche l'Ufficio parlamentare di bilancio ci dice chiaramente di guardare con attenzione tali dati, quindi ci mette in guardia soprattutto su questa relazione.

Sembra un paradosso: in un momento difficile per l'economia, il Governo che fa? Aumenta la pressione fiscale. *(Applausi)*. È un dato, come dicevo, inconfutabile. In questo momento particolare, ancora una volta il Governo che fa? Illude gli italiani, promettendo una riforma fiscale, e addirittura prevede di tagliare detrazioni e deduzioni a molte famiglie italiane, colpendo con l'assegno unico soprattutto quelle del ceto medio. Diciamo di no a queste riforme, perché da sempre siamo i veri fautori della riforma fiscale, mettendovi al centro il quoziente familiare e le famiglie, che sono importanti, per far recuperare quello che dev'essere oggi il valore

Come fate a promettere riforme fiscali, quando agli italiani oggi chiedete di pagare le tasse, comprese quelle pregresse? Siamo il Paese con la più bassa competitività fiscale. Non di secondo piano è la questione che riguarda tutti i disegni di legge collegati alla NADEF: ne sono previsti 22 nella Nota che adesso presentate; ne erano previsti 19 nella precedente.

che avete oggi di passare da annunci eclatanti a provvedimenti efficaci e concreti per il Paese. Per questo e per tanti altri motivi, che in tutti questi mesi abbiamo

Della nostra esistenza, delle opposizioni e del richiamo alle opposizioni vi ricordate soltanto quando i numeri sono ballerini. Mi dispiace, ma questa volta non caschiamo in alcun inganno. Lo ribadisco: la nostra responsabilità è solo e soltanto nei confronti del Paese e non cambiamo

Sullo scostamento da parte del Gruppo parlamentare Forza Italia non ci sarà alcun aiutino. Annuncio pertanto il voto di astensione.

responsabilità; partecipare alle soluzioni; mettiamoci insieme per fare un pezzo di strada.

Prendiamo atto che, invece, l'impegno della maggioranza e del Governo è stato quello di cercare dei responsabili, che potessero portare la maggioranza ad avere oltre 161 voti.

è stato però quello di cancellare la *flat tax* fino a 100.000 euro e di modificare quella fino a 65.000 euro, mettendo nuovi paletti, per partite IVA, artigiani e professionisti. Il secondo atto, che abbiamo visto pochi giorni fa, è stato quello di cancellare i decreti Salvini.

Se dobbiamo unire il Paese, dobbiamo anche fare un percorso culturale che vada in questa direzione. Se la logica è «cancelliamo Salvini», allora viene veramente difficile pensare che si possa trovare anche solo per un pezzo di strada, senatore Errani, un po' di convergenza.

ripeto - magari abbiamo sbagliato tutto noi e dovevamo cambiare atteggiamento. Sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,

sicuramente negativo: a parte che le previsioni delle note di aggiornamento del Documento di economia e finanza - lo sa bene il senatore Monti - non ci hanno mai preso negli ultimi quindici

a noi è dispiaciuto tanto leggere nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, nella tabella a pagina 59, che la pressione fiscale l'anno prossimo crescerà

0,1 in più. Però è un dato oggettivo: secondo la vostra Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza le tasse aumenteranno. Questo è quello che avete scritto. *(Applausi)*.

quello incarnato dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che doveva essere vicino alle aziende, alle famiglie e ai territori, vota una Nota di aggiornamento che va esattamente nella direzione opposta.

un *lockdown*, quelli notturni resteranno chiusi non si sa fino a quando, altri chiuderanno prima; ci saranno meno introiti e c'è gente che rischia il posto di lavoro. Tutte queste previsioni non sono contenute nella Nota. Come facciamo a votare a favore di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza che non tiene conto di questi aspetti fondamentali per il futuro del Paese? Sono argomenti sui quali, secondo noi, bisognava assolutamente dare una risposta chiara. Poi,

Avremmo preferito usare i soldi derivanti dallo scostamento per ridurre la tassazione. Questo accordo politico si poteva fare tra maggioranza e minoranza, anche perché, ve lo diciamo adesso, nella situazione di incertezza cui andiamo incontro in futuro,

Grazie, presidente

del Capogruppo e presidente Romeo, sul fatto che possano esserci pericoli, da qui alla fine dell'anno, per i lavoratori. In realtà, vorrei ricordare a loro e al presidente Romeo che la cassa integrazione c'è ed è stata confermata fino alla fine dell'anno: quindi, per fortuna, su questo aspetto non dovremmo avere problemi e veramente vorrei rincuorare tutti. È inutile infatti aggiungere allarme alla situazione già emergenziale che stiamo vivendo di giorno in giorno. Abbiamo letto in questo istante il dato di oggi: 7.322 nuovi casi. È molto

che sono guariti e sono tornati a lavorare tra noi; hanno avuto anche l'intelligenza e l'onestà intellettuale di avvertirci subito, quando si sono accorti di essere malati, in modo da mettere tutti nelle condizioni di correre ai ripari, se necessario.

mentre noi pativamo, per averne di molto più elevati, che appesantivano la nostra economia. Ora siamo quasi del tutto allineati e questo è sicuramente un grandissimo vantaggio per guardare al futuro. Detto questo, però, dobbiamo riconoscere che

grazie a tutto sufficiente, torneremo in quest'Aula e, come abbiamo fatto per altri provvedimenti, voteremo un altro scostamento. Lo abbiamo fatto e siamo riusciti a fare grandi cose con il decreto aprile, con il decreto crescita e con il decreto agosto. Continueremo su questa strada, perché siamo riusciti a dare benefici a moltissime famiglie e aziende. Certo, forse qualcuno è rimasto indietro e su questo dovremmo concentrarci effettivamente, perché, ogni volta che variamo una manovra, c'è sempre qualcuno che purtroppo rimane escluso. Ebbene, dovremmo concentrarci di più ed è questa la preghiera che faccio al Governo: riuscire a creare misure il più possibile universali, in modo da in modo da comprendere tutti. Mi riferisco ai vari *bonus* e alle varie misure. Purtroppo, ogni tanto, c'è qualcuno che rimane scontento, ma dobbiamo intervenire adesso, perché le possibilità ci sono: abbiamo la legge di bilancio davanti e, quindi, cerchiamo di fare effettivamente cose che servano.

sostegno, perché non possiamo perdere l'industria del turismo, che frutta il 17 per cento del PIL. Effettivamente, qualcosa in più da questo punto di vista va fatto e sono sicuro che il nostro Governo lo farà, ce lo porterà in Aula e lo voteremo. Con riferimento ad

se hanno bisogno di un'integrazione per pagare l'affitto, va garantita in misura universale, anche in questo caso, a seconda delle perdite che hanno avuto. Una volta per tutte, perché non stabiliamo che una parte ce la mette lo Stato, una parte continua a pagarla l'affittuario e una terza parte la mette il proprietario? volta per tutte, così riusciamo lentamente a tornare a una situazione di normalità. Non possiamo non pensare a chi sta peggio: i portatori di disabilità, i *care giver* e le loro famiglie. (*Applausi*). Sono le persone a cui dobbiamo fare riferimento. Nella prossima legge di bilancio, vi prego di fare il possibile per fare qualcosa

può essere migliorata con alcune cose che abbiamo già approvato nel codice della crisi d'impresa, che agevolano le procedure per il sovraindebitamento. Dobbiamo anticiparle, perché entreranno in vigore ad agosto del 2021: anticipiamo adesso le norme sul sovraindebitamento per le famiglie e riusciremo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

tutto

Onorevoli colleghi, comunico che è pervenuta, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, una proposta di questione pregiudiziale in ordine al disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in materia di proroga delle misure di contrasto del Covid-19.

Signor Presidente, l'alluvione del 2 ottobre ha spazzato via alcuni tratti di un'arteria viabile fondamentale per il collegamento tra Italia e Francia: la strada statale 20 del Colle di Tenda. Alcuni tratti di strada sono completamente inagibili e, purtroppo, anche il traforo è stato gravemente danneggiato. Quei 3.182 metri di galleria, che dal 1882 collegano la Valle Vermenagna alla Valle Roya (che in quel periodo, lo ricordo, era ancora italiana), restano tuttora inagibili. Il maltempo si è portato via anche una cinquantina di metri della strada che scende verso la Francia, a pochi metri dall'imbocco della galleria. Al posto dell'asfalto ora c'è una voragine e i tornanti a scendere sono a rischio di pericolosi e drammatici cedimenti. Sul versante italiano fango e detriti hanno reso inagibile il cantiere in corso per la costruzione della seconda canna del traforo del Tenda: uno stop che farà slittare ancora una volta chissà per quanto tempo, la fine dei lavori per il raddoppio previsti per la metà del 2024. Ricordo che questo traforo era stato ideato a partire dal 31 luglio 2001. Sono passati esattamente vent'anni e questa seconda canna non è ancora stata realizzata. Pertanto, facciamo riferimento a quello che è un problema... Nel frattempo, nel 2017 cinque sindaci francesi hanno vietato il traffico dei mezzi al di sopra delle 19 tonnellate nei Comuni francesi, con ciò determinando un blocco unilaterale verso i trasportatori e le aziende italiane che si aggiunge al danno di questi ultimi tempi dovuto all'alluvione del 2 ottobre scorso. Questo divieto è ancora in corso, con la conseguenza che la logistica deve transitare per l'autostrada o altri colli che non sono per niente comodi. Noi chiediamo al presidente del Consiglio Conte, al ministro De Micheli e all'ANAS di affrontare subito questo problema viario enorme che sta incidendo negativamente sulle imprese, sulle famiglie, sui trasporti, sulla logistica e sul turismo delle Regioni Piemonte e Liguria. una storia infinita, che ha bisogno di una soluzione immediata. Alla luce, poi, di queste fantomatiche risorse che dovrebbero arrivare, si prega fin d'ora di destinare quelle che servono a questa importantissima arteria. *(Applausi)*.

questo mio intervento è finalizzato a denunciare un'intricata vicenda relativa al riassetto delle attività del gruppo Auchan attraverso l'acquisizione da parte di Conad. di una vicenda che si è arricchita di un nuovo preoccupante capitolo che sta giungendo al culmine proprio in questi giorni e che rischia di precipitare nel disinteresse generale. Poco si dice, infatti, e nulla si sa del destino di 127 dipendenti della cooperativa General solution service, con sede legale a Lavello, divenuti - loro malgrado - un danno collaterale della partita milionaria dei supermercati che da mesi tiene con il fiato sospeso migliaia di lavoratori nel nostro Paese. Il 30 ottobre prossimo scadrà il loro contratto, che l'azienda lucana aveva legato a filo doppio con l'attività di movimentazione delle merci svolta per conto del colosso francese. Il punto è proprio questo: la necessità di fare chiarezza all'interno del complicato sistema di appalti e subappalti che ha generato quelle commesse in procinto di venir meno. Solo così sarà possibile delineare da parte dei Ministeri competenti e delle parti sociali le corrette, ma soprattutto tempestive, procedure di tutela da innescare a vantaggio dei dipendenti di Lavello e soprattutto delle loro famiglie.

avviando un'operazione trasparenza che scongiuri il rischio di creare angoli ciechi dove i lavoratori dell'indotto si ritroverebbero soli e senza via d'uscita. *(Applausi)*.

per l'attestato d'onore di Alfiere della Repubblica che ha voluto conferire, su proposta del presidente della Società italiana di pediatria, professor Villani, al giovane Sebastiano Mattia Indorato, di sedici anni. La prestigiosa onorificenza è riconosciuta dal Capo dello Stato a giovani che si sono contraddistinti per azioni coraggiose e solidali e che rappresentano modelli positivi di cittadinanza. Mattia, siciliano della Provincia di Caltanissetta, da anni si prende cura del fratellino più piccolo gravemente malato perché affetto da una malattia rara, una grave forma di encefalopatia epilettica, che necessita di cure intensive e di assistenza continuativa, mostrando estrema disponibilità e generosità fuori dal comune nell'aiutare la sua famiglia in difficoltà a fronteggiare la grave malattia e la sua difficile, complessa e quotidiana gestione, il tutto con profonda dedizione, giorno dopo giorno, spesso con rinunce silenziose alle normali attività ricreative e di svago, come le uscite con gli amici, proprie di un adolescente. Questo riconoscimento idealmente rappresenta un attestato di ringraziamento simbolico esteso a tutti i fratelli e le sorelle delle tante famiglie che, come quella di Mattia, vivono e convivono con il problema della disabilità, a garantire, pur tra enormi difficoltà, la migliore qualità di vita ai cittadini più fragili del nostro Paese. A loro Mattia ha dedicato, con spirito di altruismo e di solidarietà, l'onorificenza ricevuta, dichiarando semplicemente: «Mi piacerebbe fare qualcosa per aiutare altre persone che si trovano nella stessa situazione della mia famiglia».

e vera del nostro presente e la speranza del nostro futuro.